L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

su questa realtà, vorrei sapere che cosa intende fare e come intende applicarla il Governo. Quindi, chiedo formalmente se è possibile che il Ministro venga a riferire

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

essendo il relatore di questo provvedimento, che pare banale, ma banale non è. Vorrei rassegnarvi alcune considerazioni. La prima è questa: già mi fa piacere

di vicinanza e di solidarietà verso i nostri connazionali che vivono, operano e lavorano all'estero. È un segno di vicinanza che è bello venga da questo Senato, visto che da parlamentari rappresentiamo l'Italia tutta e che l'Italia tutta è prima di tutto un concetto spirituale. L'Italia non è soltanto quello che è dentro i nostri confini, l'Italia non è soltanto i nostri monumenti e le nostre opere d'arte, l'Italia non è soltanto tutto ciò che è materiale, ma anche molto di ciò che è immateriale: la lingua bellissima che parliamo, i valori spirituali che ci sono trasmessi attraverso le generazioni. L'Italia vive anche lontano da qui, perché esiste un'altra Italia: sei milioni e più di italiani sparsi in ogni Continente sono italiani che vivono, che lavorano, che testimoniano la loro italianità e lo fanno producendo, inventando, ideando, creando. Ci sono italiani che ce l'hanno fatta e che sono diventati grandi capitani di industria, grandi ricercatori, legislatori, legislatori, presidenti, uomini illustri del mondo; e ci sono tanti italiani che magari non ce l'hanno fatta e che vivono male, ci sono tanti italiani in difficoltà in tanti Paesi del mondo. Ma è un universo che in qualche modo rispecchia questa italianità diffusa e bellissima ed è giusto che noi facciamo sentire loro la nostra vicinanza. Questa italianità è in fondo una sorta di grande famiglia, è un po' la Patria del cuore, come ci insegnò Mazzini.

tutto ciò. Di cosa parliamo? Sono previste delle disposizioni per il finanziamento e nuovi interventi rivolti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Debbo dire che questa proposta di legge arriva dalla Camera, ma origina da una proposta dell'onorevole Toni Ricciardi del Partito Democratico (che tra l'altro è su in tribuna), meritevole di aver voluto questa legge.

empiricamente verificato (essendo un italiano all'estero) come una delle prime e quasi banali cose che chiede un italiano all'estero è avere il proprio passaporto. Un italiano all'estero, come dicevo, non sempre ce l'ha fatta, non sempre vive bene e ha spesso l'ansia di tornare a casa. Noi abbiamo all'estero italiani di vecchia generazione e italiani di nuova generazione, generazione, emigranti vecchi ed emigranti nuovi, ma, come per tutti gli emigranti, la nostalgia della casa, il voler ritornare un giorno a casa è un dato fondamentale. E la prima cosa che ti serve per tornare a casa è il passaporto. Ebbene, voi dovete sapere che le nostre strutture consolari, pur con il lavoro indefesso che svolgono, non sempre ce la fanno; spesso, anzi, non sono in grado di rispondere alle richieste. Un italiano che vuole tornare vuole tornare in Italia dall'estero, se sta in una sede fortunata, quando richiede il rinnovo del passaporto se la cava in due settimane. Ma se va male, possono passare sei, otto, dieci mesi.

il cittadino che non riesce ad avere il documento in tempi ragionevoli ripiega su altre soluzioni, ad esempio, un secondo passaporto (se in possesso di doppia cittadinanza), oppure la richiesta del passaporto in Italia, oppure rinuncia al viaggio, o rinuncia allo spostamento in aereo e viene attraverso il confine terrestre, che di solito è più facile da passare. La domanda inevasa che cosa fa percepire? Dà una percezione di abbandono da parte della Madrepatria sostanzialmente, e causa tra l'altro un disservizio grave,

per le carte di identità elettroniche e per mille altri documenti o questioni che riguardano un consolato. Io, che di queste cose mi occupo, vi potrei raccontare ad esempio la settimana scorsa, quando ero in Marocco, ho appreso che il solo consolato di Marrakech, con tre persone, deve gestire una richiesta di 150 atti al giorno, tra passaporti, richieste di visti e quant'altro: è semplicemente impossibile, quindi è lavoro che si accumula.

Sono inascoltati da tempo. Questa notte mi hanno scritto dal Brasile, dove continua invece un'altra questione molto strana, quella delle prenotazioni per avere i passaporti,

Il disegno di legge stabilisce che sia stanziato un fondo, che sarà di quattro milioni annui, diretto a finanziare le strutture consolari perché siano adibite a questo tipo di lavori. una dotazione pari a quattro milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinata al finanziamento di interventi per il rafforzamento dei servizi consolari in favore di cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti, compresi quelli relativi al rilascio di passaporti. Nel medesimo comma viene altresì previsto che le risorse del fondo siano ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero di passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente. Il secondo comma stabilisce che, entro il 31 di marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, nel sito Internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia pubblicata un'apposita relazione che contenga i dati aggregati relativi all'utilizzo delle somme del fondo. il terzo comma reca la copertura finanziaria del provvedimento e dispone, come dicevo, che gli oneri derivanti dalla legge saranno pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. 2025. Ho terminato l'illustrazione, alla quale tenevo. Vi ho fatto perdere qualche minuto in più, perché qualcuno mi invitava a concludere, però dico che, quando siamo in questo Parlamento e discutiamo di cose serie, si può anche perdere qualche minuto in più e sono fiero di averlo perso.

ai nostri consolati, che sono in grave difficoltà; il nostro corpo diplomatico in genere è in grave difficoltà, le nostre rappresentanze diplomatiche coprono anche sedi molto importanti con un numero di diplomatici che sono spesso la metà o un terzo di quelli impiegati da Paesi grandi come l'Italia. ogni qualvolta possiamo dare una mano ai nostri diplomatici che fanno un lavoro straordinario - devo dirlo - con una grande reputazione intorno al mondo, credo che non ci possa essere esitazione e che si debba votare in quella direzione. necessario che i nostri italiani all'estero possano essere assistiti dai nostri consolati in modo adeguato, quindi dare maggiori fondi ai ai nostri consolati all'estero è una cosa che va assolutamente fatta e dunque voteremo a favore. Detto questo, però, e avendo annunciato il voto favorevole, sarebbe secondo me miope e anche ipocrita non andare a scavare un po'

risolviamo il sintomo, quindi se abbiamo la febbre, prendiamo l'aspirina. Tuttavia, se abbiamo la febbre c'è sempre una causa e sarebbe più opportuno prendere l'antibiotico, fare in modo che la causa passi. Se leggiamo il testo del disegno di legge ci accorgiamo che i soldi che noi andiamo a stanziare servono a rafforzare servizi consolari in favore di cittadini italiani residenti e presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Ci sono molti servizi che vengono richiesti ed è giusto che la nostra rete consolare li fornisca ai nostri concittadini; tuttavia, come giustamente diceva anche il relatore Menia, sappiamo benissimo che che a mettere in difficoltà la rete dei nostri consolati sono i passaporti, che sono un problema anche per gli italiani che vivono in Italia: chiedere un passaporto nel nostro Paese è una sfida all'Ok Corral, cioè di solito di solito bisogna avere un'urgenza che non si può fermare, perché altrimenti bisogna aspettare dei mesi (quando va bene). Tuttavia, la ragione per la quale i nostri consolati sono in difficoltà dobbiamo chiamarla con un nome e un cognome ed è l'assurda legge sulla cittadinanza che abbiamo in Italia, che stabilisce che è cittadino italiano chiunque abbia un avo,

con parole molto alte, descriveva l'amore dei nostri connazionali per la nostra lingua; tuttavia, io che ho frequentato i consolati italiani all'estero, avendo vissuto molto tempo all'estero, posso assicurare al collega Menia che nei nostri consolati va molta gente che non parla neanche una parola di italiano, perché l'Italia non l'ha vista manco col cannocchiale. Si tratta di persone che sono non solo magari discendenti di gente che è andata via nell'Ottocento, ma sono anche i loro coniugi, per cui per esempio i figli dei loro figli sono persone che con l'Italia non hanno alcuna relazione, zero assoluto, ma hanno diritto a un passaporto italiano.

(quindi, gente che è stata residente in Italia per dieci anni, 59.000 minori figli di questi immigrati), quindi 169.000 residenze.

parlano italiano, pagano le tasse in Italia, collaborano e contribuiscono alla prosperità del nostro Paese: giovani, anziani, persone che vivono in mezzo a noi, che gestiscono le nostre imprese, che lavorano in mezzo a noi, che vanno a scuola. Ebbene, queste persone fanno una fatica enorme a ottenere un passaporto, mentre siamo costretti a dare più soldi ai nostri consolati perché non ce la fanno più: se le cose stanno così, non solo non ce la fanno i consolati, non ce la fanno neanche i nostri tribunali. Il presidente del tribunale di Venezia, il dottor Laganà, ha ricordato che a Venezia ci sono 25.000 ricorsi

che ha 3.000 residenti e 1.700 residenti all'estero, dove ci sono 500 pratiche che aspettano e il TAR del Veneto ha dato

benissimo, allora, dare più soldi ai nostri consolati, tant'è che io, entusiasticamente, insieme al mio Gruppo, voterò per sostenere il nostro corpo diplomatico, i nostri italiani all'estero, ma cerchiamo

cittadinanze per *ius sanguinis* e meno di 170.000 a persone che dimostrano la loro italianità non su base etnico-razziale, non sulla base del fatto che hanno un cromosoma

una sorta di pannicello caldo: certamente il nostro console a Mar del Plata, che è sommerso non tanto dal Mar del Plata, quanto dal mare di richieste di passaporti, non credo che ci farà granché. Penso che dobbiamo rimettere un minimo di razionalità in tutta questa discussione, ma ovviamente non sostenendo solo i nostri consoli, perché le nostre ambasciate sono ampiamente sottostaffate diplomatici fanno fatica a rappresentare un Paese importante come l'Italia, con i numeri che hanno. Abbiamo tante ambasciate importanti dove c'è un solo diplomatico, al

è solo il sintomo di una febbre che non possiamo curare con la Tachipirina, anche se so che questa maggioranza di Governo ha una grande familiarità con la Tachipirina (ce lo ha ricordato la sorella della Presidente del Consiglio).

che, per quanto ci riguarda, è un primo passo. Quanto infatti detto prima di me dal senatore Scalfarotto sulla questione della cittadinanza e sui servizi in generale, anche sul finanziamento che deve servire per dare risposte concrete ai cittadini,

Raggiungeranno presto questo numero, posto che il saldo migratorio nel 2022 è stato di circa 20.000 italiani usciti in più rispetto a quelli rientrati; 100.000 sono espatriati e 75.000 sono rientrati. Siamo di fronte a una nuova ondata, largamente, ma non solo, composta da quelli che chiamiamo i cervelli italiani. flussi in uscita che si uniscono all'antica immigrazione italiana che ha contribuito a fare prosperare le economie di molti Paesi nel mondo. Allo stesso tempo quei coraggiosi italiani all'estero hanno partecipato alla crescita di quella italiana, che ha beneficiato delle rimesse generose di chi era andato all'estero per lavorare, farsi una posizione e creare ricchezza. Sempre nel 2022 hanno acquisito la cittadinanza italiana 85.000 persone residenti all'estero. quindi di fronte a un numero di italiani all'estero che cresce di anno in anno. La rete consolare italiana è composta da 123 ambasciate, 77 consolati e 8 rappresentanze permanenti in tutto il mondo. Ecco quindi che il disegno di legge al nostro esame si pone l'obiettivo di andare incontro alle esigenze degli italiani nel mondo, non solo con un segnale di attenzione, ma con un'azione concreta per incrementare i servizi che vengono loro forniti. La *ratio* del provvedimento è quindi assolutamente in linea con la grande considerazione dimostrata dal ministro Antonio Tajani verso le sedi estere, fin dal suo insediamento alla Farnesina. Si tratta di un'attenzione che si è manifestata potenziando la struttura diplomatica e consolare italiana attraverso nuove assunzioni. proposta è certamente da apprezzare perché mette in campo nuove risorse per rafforzare i servizi consolari per gli italiani all'estero. È un disegno di legge di iniziativa delle opposizioni, messo a punto dal lavoro della Camera, in accordo con il ministro Tajani e il Ministero da lui sapientemente guidato. Per queste buone ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. Signor Presidente, colleghi, consegnerò il testo dell'intervento e mi permetto di fare solo due considerazioni, collegandomi a quanto detto sia dal relatore che dal senatore Scalfarotto poc'anzi, un'ultima considerazione su quanto prevede una parte del disegno di legge. Credo che dare quattro milioni ai consolati sia cosa buona e giusta, anzi sarebbe da darne di più. Mi chiedo se il criterio utilizzato nel disegno di legge sia quello più corretto. Le risorse del fondo saranno ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati l'anno precedente. Come ha fatto notare il relatore Menia, abbiamo

interinale proprio a supporto di quegli uffici che meno degli altri possono contribuire a sveltire le pratiche. Inoltre, credo che tutti noi abbiamo nelle nostre caselle *e-mail* segnalazioni,

segnalazioni, perché si parla di migliaia di euro per un visto. Ora, io sono assolutamente convinto che il personale dei consolati sia formato da persone oneste. Ma il meccanismo che si è creato permette a malintenzionati, se non delinquenti, di lucrare sulla pelle delle persone che chiedono banalmente un servizio cui hanno diritto. Io credo che occorra rivedere tutto il meccanismo.

in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Lo scopo dell'intervento normativo è di rafforzare la capacità della nostra rete consolare, di evadere in maniera più rapida le domande di passaporto e di altri documenti di identità.

In primo luogo, per la prima volta si rende strutturale e si segue un *iter* ordinario

gli eletti all'estero cercavano di ottenere attenzione. Invece, per la prima volta, riusciamo a costruire un intervento strutturale in via ordinaria, ed è sicuramente un passo in avanti. C'è poi una seconda motivazione, lo facciamo con uno spirito *bipartisan*. Ho apprezzato molto le parole del relatore, il vice presidente Menia, che ha riconosciuto

Vero è - come ha detto il collega Scalfarotto - che noi dobbiamo bilanciare un'attenzione al tema della cittadinanza, che noi diamo a persone che abbiano un vero legame con l'Italia, col nostro territorio culturale e professionale di origine, che è anche utile nel rapporto fra i diversi Stati, insieme a chi decide di avere qui la sede dei propri affetti e del proprio di rispettare le leggi e di pagare le tasse e a coloro che vanno a scuola con i nostri figli. Noi non li possiamo più far aspettare. Dobbiamo estendere la cittadinanza a chi ha deciso di avere qui la sede della propria della però, stiamo parlando d'altro. Stiamo parlando della ventunesima regione del nostro Paese: quasi sette milioni di donne e di uomini iscritti all'AIRE. E attenzione ad essere fuorvianti, perché il 65 per cento degli iscritti all'AIRE sta in Europa ed è emigrazione consolidata. Parliamo, però, anche di una nuova mobilità, di nuovi flussi migratori, di giovani che vanno all'estero per inseguire un'occasione professionale, per costruirsi una famiglia. E noi a questi italiani all'estero dobbiamo dare servizi e dobbiamo tutelarli. Molto spesso si sottovaluta il fatto che i consolati all'estero sono il luogo in cui i nostri cittadini trovano le risposte che trovano nei Comuni. Spesso noi raccontiamo, giustamente, come i Comuni siano il livello più vicino ai cittadini e diano risposte nel quotidiano. All'estero quelle realtà sono i consolati e molto spesso i consolati non sono messi nella condizione, perché non hanno le risorse, di rispondere a quei bisogni. *(Applausi)*. Ecco perché ha valore questo provvedimento, che poteva essere più ampio,

agli altri servizi. È comunque un segnale per la comunità all'estero. Si parte dai passaporti, per i quali spesso le comunità all'estero devono aspettare anche sei mesi, con liste di attesa enormi, per estendere anche ad altri servizi. Noi vorremmo che fosse così, che questo diventasse

è un provvedimento che, in futuro, si autoalimenterà. Mediamente, noi emettiamo circa 500.000 nuovi passaporti,

tra i diversi Paesi, tra le comunità di origine e le comunità dove sono andati a lavorare e a portare ricchezza. Ecco perché, come Partito Democratico, anche con una punta di orgoglio, salutiamo positivamente questo provvedimento, che fa fare un passo avanti nella tutela e nella difesa delle nostre comunità di eletti all'estero.

il provvedimento in esame è particolarmente importante. Come ha ricordato bene chi mi ha preceduto, è importante per i nostri connazionali all'estero ed è importante per la nostra immagine nel mondo. La nostra comunità, ben seguita, è una comunità che ben ci rappresenta. Quindi, i nostri concittadini che riescono ad avere risposte dai nostri uffici consolari sono concittadini che meglio rappresentano l'Italia. Questo è un atto non solo doveroso, ma è anche urgente e necessario. Aumentare l'organico nei nostri consolati, soprattutto amministrativo, è utile per velocizzare

problemi degli italiani. Con questa maggioranza e con il Governo Meloni l'Italia e gli italiani ci rivedono protagonisti nel mondo. Era ora. Avere consolati che lavorano meglio significa avere illustri cittadini

che aveva lanciato un'ombra su un possibile Governo di destra, che si sarebbe chiuso nelle proprie grigie stanze e non avrebbe mai avuto la capacità di dialogare con Nazioni, Stati e *leader* mondiali come quelli americano, inglese, indiano, cinese o giapponese, con territori aspri e problematici come l'Africa. Ha sempre pensato che non saremmo mai neanche riusciti a uscire sul balcone per esprimere la felicità di aver finalmente risolto il problema della povertà. Si è invece ritrovato, dopo soli due

È proprio nelle ultime ore che possiamo vedere quanto questo Governo stia riuscendo a stare nella

l'auspicio di riuscire a fare sempre meglio nei prossimi tre anni, collaborando anche con le minoranze, laddove ci siano proposte che possiamo ampiamente sposare come questa, voglio fare gli auguri da parte di Fratelli d'Italia al collega Raffaele Fitto *(Applausi)*, che proprio nella serata di ieri ha ricevuto ufficialmente l'incarico. Questa è una vittoria - lo ribadisco - non solo per un Governo, ma è la vittoria di una Nazione, la vittoria dell'Italia, la vittoria degli italiani. Ho cercato, grazie alla richiesta del collega Boccia, di ridurre il mio intervento al minimo indispensabile, senza mai dimenticare che anche in un provvedimento come questo occorre ricordare cosa si è fatto e cosa si farà. Ovviamente esprimo il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

La relatrice, senatrice Spinelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Signor Presidente, prima di svolgere la relazione, permettetemi di esprimere la massima solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie delle vittime di eventi derivanti da cedimenti di infrastrutture. del Governo, onorevoli colleghi, oggi approviamo il testo unificato, approvato in sede redigente dalla 1a Commissione affari costituzionali lo scorso 9 ottobre. Il tema è importante e delicato: parliamo appunto di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali e autostradali di rilievo nazionale, partendo dalla tragedia del 14 agosto 2018 a Genova. Abbiamo ascoltato le istanze presentate dal Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi e, insieme a tutti i membri della Commissione guidata dal presidente Alberto Balboni, abbiamo lavorato a un testo unificato. Come relatrice ringrazio i firmatari dei disegni di legge, la senatrice Minasi, il senatore Basso. E desidero rimarcare altresì che entrambi i disegni di legge nn. 794 e 868 sono stati sottoscritti dalla senatrice Paita, che ringrazio per l'impegno e il sostegno che ha sempre garantito *(Applausi)* anche da Presidente della Commissione trasporti della Camera nella scorsa legislatura, affinché avvenisse un esame celere e approfondito del provvedimento stesso. Il disegno di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione. Gli eventi dannosi saranno individuati da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di quelli che si sono verificati nell'arco temporale dal 13 agosto 2018 alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità di individuare con successivi decreti altri eventi che si sono verificati in seguito all'entrata in vigore della legge in esame. L'articolo 2 prevede il fondo per iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime. Tale fondo ha una dotazione di sette milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni per l'anno a decorrere dal 2026. Viene stabilito così l'ordine che individua i membri delle famiglie beneficiarie e si precisa che, in presenza di figli a carico delle vittime, nati da rapporti di convivenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76 del 2016, la speciale elargizione viene corrisposta anche al convivente superstite, secondo l'ordine di priorità previsto per le ipotesi in cui vi siano un coniuge superstite e i figli a carico. Oltre a questa totale elargizione si prevede, con decreto del Presidente, che possano essere riservate, nei limiti chiaramente delle risorse di fondo, ulteriori iniziative di solidarietà sociale. Nell'articolo 3 sono specificati beneficiari. L'articolo 4 individua lo strumento deputato alla ricognizione degli eventi. L'articolo 5 prevede la possibilità di accedere alle assunzioni dirette da parte dello Stato, un diritto di collocamento obbligatorio valido per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3. L'articolo 6 prevede la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi, per ogni anno di scuola primaria e secondaria di primo o secondo grado o corso universitario; si tratta di borse di studio pari a 100.000 euro, a decorrere dal 2025, esentate da imposizione fiscale. L'articolo 7 prevede misure a favore dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia deceduti nell'evento. L'articolo 8 individua la copertura finanziaria e l'articolo 9 l'entrata in vigore del provvedimento. Il principio su cui tali disposizioni si fondano è quello della solidarietà sociale. Questo intervento dello Stato costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria. Presidente, vorrei ringraziare il Senato per aver portato in Aula questa proposta di legge, che vede che vede tutte le forze politiche concordi. Credo che sia un bel segnale per il Paese e soprattutto per le vittime del disastro che c'è stato a Genova nel 2018, ma anche per tutte quelle che speriamo non ci siano mai, ma che in qualche modo sono relative a manufatti, viadotti o opere sul territorio nazionale che non vengono gestiti o mantenuti e che rischiano rischiano di creare dei problemi. Credo che il 2018 abbia segnato una svolta sulle norme di edificazione e creazione delle nuove infrastrutture. In questo momento abbiamo anche il cambiamento climatico e, quindi, dobbiamo creare norme che rendano ancora più resilienti le nostre infrastrutture. Bisogna in qualche modo far sentire i nostri cittadini protetti, in una situazione di cambiamento e di rinnovamento del sistema infrastrutturale nazionale. Credo che in questo caso le forze politiche e il Senato tutto abbiano dimostrato una particolare attenzione e abbiano dato risposta a un'esigenza che ci trasciniamo dal 2018 e che finalmente oggi

Signor Presidente, voglio essere molto chiara: questa è una giornata importante per il Parlamento, anche se dalle dalle voci e dalla disattenzione potrebbe non sembrarlo. In realtà lo è, perché considero l'atto di oggi il completamento di un percorso di ricostruzione di fondamentali rispetto a come lo Stato deve occuparsi e rapportarsi con il tema delle concessioni. iniziato con la redazione del decreto-legge Genova e poi, a seguito, con tutta la reazione che c'è stata in merito a quell'enorme, immane tragedia che ha portato quarantatré vittime e che ha sancito un momento veramente molto complicato per la vita del Paese e sicuramente per la vita della regione Liguria. Per queste ragioni, voglio innanzitutto richiamare l'attenzione di tutti voi sull'esigenza di ringraziare una persona che in questi anni non ha mai smesso

alla sua capacità di reazione, alla dignità con la quale ha voluto portare avanti una battaglia non solo per le vittime del Ponte Morandi, ma per tutte le vittime dell'incuria e dell'assenza di manutenzione nel nostro Paese. nel nostro Paese. Il sottosegretario Rixi va altresì ringraziato, perché ha fatto un lavoro di cucitura che però non è partito da questa legislatura: in realtà la richiesta da parte del Comitato

è venuta nella Commissione trasporti della Camera e nella Commissione ambiente e infrastrutture della Camera, alle Presidenti di allora, ossia la sottoscritta e Alessia Rotta, che voglio ricordare per il lavoro importante che in quel caso aveva fatto. Da lì erano partite le prime iniziative legislative, che poi sono la base e il supporto del lavoro di oggi. Quando è terminata la precedente legislatura non si era ancora arrivati all'approvazione definitiva di questo disegno di legge, e c'erano stati anche dei rilievi di carattere formale per i quali era giusto intervenire con delle modifiche puntuali. A quelle modifiche hanno lavorato il sottosegretario Rixi, che appunto ringraziamo per l'impegno, ma anche il ministro Salvini. Oggi pomeriggio nel *question time* sarò durissima con il ministro Salvini, ma, siccome sono una donna delle istituzioni, voglio riconoscere che su questa vicenda il ministro Salvini ha fatto un lavoro di tessitura: ha riunito tutti i firmatari dei progetti di legge; lo ha fatto in una riunione pubblica; abbiamo dato in quell'occasione l'assenso a lavorare a un testo unitario che la relatrice richiamava, su cui sono state apposte tutte le nostre firme e tutte le nostre proposte. inoltre che il ministro Salvini ha rapidamente fatto in modo che il Governo sostenesse questa iniziativa. Quindi, istituzionalmente oggi stiamo facendo una cosa buona e doverosa,

però, che sia anche l'occasione per dirsi delle cose con franchezza su ciò che, invece, ancora non va. La vicenda del Ponte Morandi segna un discrimine, perché perché è crollata un'infrastruttura che era stata data in concessione ad un privato e che, a causa dell'assenza di manutenzione ora non si può ancora dire definitivamente, perché è ancora in corso un processo, ma sicuramente anche a causa di quella assenza di manutenzione è crollata, determinando la perdita di vite di cui parlavo prima. Quella vicenda, per chi si ricorda, aprì un dibattito nel nostro Paese: il solito dibattito in cui si deve trovare il responsabile immediato di tutto quello che era stato fatto o che non era stato fatto. E ricordo un dibattito sbagliato: per esempio il MoVimento 5 Stelle aveva messo in atto una caccia alle streghe nei confronti dell'ex ministro Graziano Delrio, che io invece desidero ringraziare, perché ha lavorato benissimo da Ministro e aveva fatto delle cose importanti. Quello che invece da questa vicenda ancora non si è potuto elaborare fino in fondo in termini di nuova iniziativa è il fatto che, se andiamo a vedere bene, un miglioramento reale del potere di controllo del Ministero nei confronti dei concessionari ancora non c'è. E lo dobbiamo dire con nettezza, perché purtroppo correremo dei rischi, senza la capacità di avere come Ministero una postura giusta nei confronti di beni che - lo ripeto - sono dati in concessioni, non sono regalati al privato; sono dati in concessione e, quindi, hanno bisogno di una costante manutenzione, di una costante verifica sul piano degli investimenti, di una costante capacità di controllo sui temi della sicurezza, sulla messa in sicurezza delle gallerie e dei viadotti. viadotti. Solo in questo modo non solo si garantisce la sicurezza dei cittadini, ma si fa anche in modo di avere una capacità di investimento sulle opere che non sia una dispersione di risorse e di energie. Ci tengo a dire

credo che sia un valore per tutti. Ci devono essere, colleghi, dei codici unificanti in questo Parlamento, altrimenti come facciamo a progredire in termini di legislazione, se non ci riconosciamo vicendevolmente le cose buone che ha fatto Delrio, le cose buone che ha fatto Bucci, le cose buone che in questo caso hanno fatto Rixi e Salvini? Lo dico perché questa è una materia complessa, che richiede molta serietà e molto rigore. Noi abbiamo, da un lato, ricostruito un ponte che era crollato, certo non sanando la ferita di quelle morti, ma dando la dimostrazione che c'è stata una reazione da parte di una comunità

un segno importante per non dimenticare, ma anche un monito al Parlamento, per fare in modo che leggi e controlli avvengano in forme diverse. Si è emanato un provvedimento che ha aiutato in parte la comunità: luci e ombre, ma sicuramente ci sono anche delle luci in quel provvedimento. Oggi abbiamo un quarto atto da fare, e cioè avere una discussione franca e il più possibile anche proficua sul fatto che noi dobbiamo avere una capacità di controllo su tutte le concessioni (ferroviarie, portuali, stradali, autostradali), in modo tale che il margine di controllo, di verifica e di rischio sia il più possibile ridotto. Per fare questo, certo bisognerebbe andare

pur avendo un compito molto importante, che è quello di sancire il principio che la gestione del privato non è il male, ma che il pubblico non può ritrarsi e far fare solo al privato,

oggi tenevo a intervenire: non solo perché quella è stata una vicenda che ha ferito moltissimo la mia comunità, ma perché penso che sia emblematica di di un dramma e di un dolore, ma anche di capacità di ascolto di chi quel dolore l'ha provato ed è stato capace di reagire con varie iniziative che ho cercato di descrivere, delle quali dobbiamo dare a tutti, nome per nome,

ad essere dimenticate, ma ad affievolirsi nel ricordo, spero che questa vicenda rimanga invece molto nitida nella memoria di ognuno di noi, perché purtroppo se dovessi rispondere alla domanda se oggi dal punto di vista della sicurezza siamo tranquilli su ogni viadotto, su ogni ponte, su ogni galleria, non potrei dare una risposta positiva. È per questo che dobbiamo lavorare e dobbiamo farlo restando il più possibile coesi su una materia che - lo ripeto - non può essere una bandiera per nessuno, ma deve essere un impegno per tutti.

perché di fronte alla tragedia del ponte Morandi il Parlamento oggi definisce lo

di un solo caso, ma questa definizione è estensiva; il cantiere è l'insieme dello stato di incuria che esiste nel nostro Paese

di come calpestiamo in modo sbagliato il suolo anziché conservarlo. In sostanza vorrei sottolineare che in questo caso lo Stato diventa il responsabile e quindi ha il compito e - direi di intervenire su tutto questo. Ciò vorrebbe dire che questa è una definizione di *status*, ma adesso arrivano

credo che vadano stanziate risorse non per grandi opere, ma per un intervento sull'antisismicità, sul contenimento energetico, sulla questione della sicurezza stradale e dei

Grazie, senatore Magni, tutti noi abbiamo negli occhi le immagini del Ponte Morandi, che fu spaccato in due, e la montagna di macerie dopo che 250 metri di carreggiata caddero a terra nella valle del Polcevera, andando a coprire 43 vite innocenti spezzate da un volo di 90 metri. Era esattamente il 14 agosto di sei anni fa. I tre consulenti esperti nominati dal giudice per le indagini preliminari nelle due perizie svolte durante gli incidenti probatori scrissero testuali frasi: «la causa scatenante il crollo è la corrosione della parte sommitale del tirante della pila 9 che ha mostrato un'evidente e gravissima forma di corrosione nella zona di attacco con l'antenna», la quale «ha avuto luogo in zone di cavità e mancata iniezione formatasi nella costruzione del ponte». «La mancanza e/o l'inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema». Se i controlli «fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente, avrebbero interrotto la catena causale e l'evento non si sarebbe verificato». Vero, noi sappiamo comunque che la giustizia sta andando avanti, ma ancora non sono stati individuati i responsabili. Tutti noi abbiamo il dovere morale di individuare i colpevoli, farli riconoscere e rispondere in questo caso alla giustizia,

responsabilità gestionale i concessionari di quel tratto autostradale ha portato ai risarcimenti da parte delle assicurazioni. Ovviamente non tutte le vittime e i loro parenti hanno però accettato gli indennizzi proposti dalle compagnie assicuratrici. Lo Stato - possiamo dire - ha prontamente reagito con decisione a quella disgrazia, che qualcuno ha definito una tragedia annunciata. Il viadotto è stato ricostruito con una procedura innovativa e anche in tempi ragionevolmente brevi. Da quel disastro, però, dobbiamo trarre insegnamento, posto che l'elenco delle infrastrutture a rischio sappiamo che purtroppo è molto lungo. Molte sono infatti quelle costruite prima del 1974, anno da cui diventa obbligatorio il rispetto delle norme antisismiche per costruire. Non c'è un elenco preciso delle opere fatiscenti, anche se sono uscite diverse stime che individuano in qualche centinaio, forse 600, le opere che oggi sono a rischio. Il Ministero delle infrastrutture ha messo in campo le linee guida che conosciamo per la classificazione e gestione del rischio, anche per valutare la sicurezza dei ponti esistenti. L'esame in Commissione ha portato alla scrittura più puntuale di un testo, che ora riguarda i benefici, a livello internazionale, in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali. L'oggetto del L'oggetto del disegno di legge, quindi, oggi rimane il risarcimento delle vittime o dei familiari delle vittime che perdono la vita in eventi dannosi. Il fondo che viene ora costituito rappresenta, quindi, una vera e propria forma di assicurazione, dotata di risorse appostate nel bilancio dello Stato. Un fondo pronto ad essere utilizzato, ma che bisogna ovviamente alimentare ogni anno, perché sappiamo benissimo che le risorse non bastano mai, quindi tutti noi dobbiamo assumerci le responsabilità nei confronti delle vittime. Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. «nel 2019 Atlantia distribuisce la bellezza di 716 milioni di euro, oltre 220 dei quali alla famiglia Benetton. Ai più alti *manager*, tra cui Giovanni Castellucci, ASPI riconosce 11 milioni di euro di premi. Alcuni fra loro sono già indagati dalla procura di Genova per reati gravissimi. Nella relazione di bilancio non viene spesa nemmeno una riga per i morti di Genova, che, evidentemente, qualcuno spera vengano presto dimenticati. Il crollo di un ponte è un evento rarissimo nella storia dell'ingegneria mondiale. Tuttavia, questa non è solo la ricostruzione di un disastro, quella del ponte Morandi è una storia italiana. Racconta di un gestore privato che si è arricchito tagliando le manutenzioni e di un controllore pubblico che non controllava. Ma soprattutto, di come sia servita una catastrofe per accorgersi che nessuno sorvegliava l'opera più a rischio del Paese. In questa storia la verità viene nascosta, i documenti falsificati, le indagini depistate, e chi compie verifiche o indaga viene trasferito. L'inchiesta apre uno squarcio su un sistema che ha consentito ai signori del casello di fare soldi a palate, lasciando deperire le infrastrutture che nel frattempo invecchiavano: la privatizzazione della rete autostradale italiana, un bene pubblico, si è rivelata un affare solo per i privati». Queste, Presidente, non sono parole mie, ma è lo stralcio di un libro che si chiama «Il crollo», del giornalista Marco Grasso, che ha raccontato la tragedia del ponte Morandi.

questa, purtroppo, è una storia italiana. Non è una storia italiana perché è successa in Italia, ma perché purtroppo evidenzia alcuni dei peggiori difetti di questo Paese. È una storia italiana perché lo Stato non ha fatto lo Stato, lo Stato, ma ha dato a un privato un bene pubblico in regime di monopolio e di fatto non ha controllato cosa questo privato facesse: il privato si controllava da solo. È una storia italiana perché racconta di un rapporto malato tra una certa finanza e una certa politica, che ha permesso che quell'evento potesse accadere e che chi aveva la concessione di quel bene beneficiasse anche di un contratto capestro, che prevedeva che, anche in caso di evento causato da dolo grave, si dovessero riconoscere tutti i mancati pedaggi, anche in caso di revoca della concessione, fino a 20 miliardi di euro. È una storia italiana perché racconta non di imprenditori, ma di "prenditori", di chi riesce ad avere, in modo miracoloso, la gestione di una tratta autostradale, di fatto non mettendoci un euro, con un'operazione a debito per sette miliardi miliardi di euro, aumenta i pedaggi e con l'aumento dei pedaggi paga un debito. Questo non è essere imprenditori, questa è un'operazione che può fare chiunque; chiunque abbia evidentemente gli amici giusti che gli consentano di farlo.

e ha devastato le loro famiglie, cui oggi noi diamo un segnale positivo. È una cosa molto bella, ancorché normale, che il Parlamento voti all'unanimità. però evidente che non andiamo a risarcire nessuno. Lo facciamo da un punto di vista economico, ma quello che è successo non prevede nessun risarcimento. Il nostro auspicio è che qualcosa del genere non possa più accadere. Quindi, al di là di questo provvedimento sacrosanto, che, lo ripeto, noi votiamo con convinzione, ciò che dobbiamo fare è adoperarci perché non succedano più cose del genere, perché non ci sia più un rapporto così profondamente sbagliato e malato tra alcuni mondi finanziari e alcuni mondi politici, perché questa perché questa è una storia drammatica che ci racconta molto bene come l'incuria e il disinteresse della politica possa portare a una soglia molto labile tra l'essere ed il non esserci. Signor Presidente, chi le parla quella mattina è passato sul ponte Morandi alle ore

Il risultato è stato che fare colazione pochi minuti prima o scegliere di passare da una parte o dall'altra, quel giorno ha condotto 43 persone verso una tragedia immane, di cui si è occupato tutto il mondo. È una ferita che non si può sanare con questo provvedimento. una ferita che non si rimarginerà mai per l'Italia ma, evidentemente, soprattutto per la città di Genova. Quindi, credo sia importante quello che approviamo oggi. Vorrei ricordare le parole di Egle Possetti, la presidente del Comitato dei parenti delle vittime, sempre citando il libro di cui parlavo prima, che dice: la forza del legame che unisce le vittime di un disastro è semplice da spiegare: è una comunità di persone che si capisce perché vive le stesse cose; una comunità che si è ritrovata insieme, suo malgrado, perché ha perso i suoi affetti e ha avuto la vita devastata. Il nostro cuore è rimasto sotto quelle macerie. Da questa esperienza, proviamo a trarre un senso: perché un fatto simile non si ripeta, perché altri non debbano subire quello che noi abbiamo subito, per cercare verità e giustizia, per provare a lasciare dopo di noi un mondo migliore.

evidentemente portati alla conclusione di mettere avanti l'interesse dei parenti delle vittime e non quello della nostra singola forza politica.

*(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signori del Governo, oggi discutiamo un disegno di legge che nasce purtroppo dal dolore, il dolore di tante persone e tante famiglie, causato da una tragedia probabilmente evitabile e dall'urgenza di garantire

l'allora vice ministro Rixi (che non era a Genova, ma in un'altra città) rientrare velocemente per accorrere ed essere di supporto nelle fasi iniziali della tragedia in cui, realmente, non si capiva l'entità dei danni e delle

Il crollo del ponte Morandi è stato una sorta di spartiacque nella storia del nostro Paese: un Paese di grandi ingegni e opere, che però ha dimostrato tutte le sue gravissime carenze nella gestione, manutenzione e vigilanza delle infrastrutture. C'è un prima e un dopo il ponte Morandi, che ci ha costretti a riflettere sulla responsabilità del sistema e ad allargare questa riflessione a tutti i casi in cui da quelle responsabilità derivino, purtroppo, conseguenze nefaste, come quelle a cui abbiamo assistito in quell'occasione. Dunque, abbiamo capito che non potevamo rimanere inerti e immobili, ma che dovevamo intervenire e lo abbiamo fatto con questo disegno di legge, che vuole dare una risposta concreta concreta e coraggiosa. Si tratta, infatti, non solo di un provvedimento tecnico, ma anche di un atto morale, sociale e istituzionale che si fa carico di sostenere le vittime degli eventi causati da cedimenti strutturali e prevenire nuove tragedie attraverso una serie di misure di controllo e responsabilità. È sufficiente soffermarsi sui punti centrali del provvedimento per capire che esso trova la sua forza e il suo presupposto nei princìpi solidaristici sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, introducendo un sistema articolato di misure a favore delle vittime e delle loro famiglie. Anzitutto, è prevista l'istituzione di un fondo di solidarietà, con una dotazione iniziale di sette milioni di euro a partire dal 2025 e 1,5 1,5 milioni di euro per gli anni successivi, per offrire un supporto economico immediato e iniziative di sostegno al reddito delle famiglie delle vittime, che ci auguriamo non si ripetano o si riducano drasticamente. Gli interventi non si limitano a un risarcimento simbolico, ma includono misure integrate che accompagnano i familiari nel superare l'emergenza e ricostruire una prospettiva di vita dignitosa. Prevediamo, poi, che i benefici economici siano cumulabili con risarcimenti privati di altra natura, compresi quelli relativi al danno non patrimoniale. che può sembrare poco incisiva, in realtà evita conflitti legali, assicurando che il supporto economico sia rapido ed efficace. Questa è un'esigenza sicuramente primaria per chi vive una tragedia di questo tipo. Vi sono poi interventi a favore dell'istruzione e della formazione. Abbiamo pensato a coloro i quali, malauguratamente, si trovino a perdere i genitori a seguito di drammi legati a cedimenti infrastrutturali, ritrovandosi così orfani all'improvviso, e che debbano essere presi sotto l'ala protettrice dello Stato e non si debbano sentire abbandonati, sommando al proprio dolore anche una penalizzazione in termini di opportunità per il futuro. Abbiamo previsto per questi soggetti borse di studio esenti da imposizione fiscale, che coprano l'intero ciclo educativo, dalla scuola primaria all'università. Sicuramente questa è una misura che, più di altre, riteniamo pregna di significato in quanto si tratta non solo di un atto di giustizia, ma anche di una piccola forma di risarcimento per chi ha subito un danno per colpe altrui. Dello stesso tenore sono il collocamento obbligatorio e il supporto lavorativo per i familiari superstiti, che avranno accesso a misure di collocamento nella pubblica amministrazione. Si tratta di un sostegno fondamentale per garantire stabilità economica e sociale alle famiglie colpite. Anche questa è una forma di risarcimento, un'opportunità veramente importante di supporto nei confronti di chi ha vissuto il dolore per una perdita che è certamente non colmabile, ma che quantomeno può essere lenito. inoltre, introduce misure specifiche per facilitare l'accesso alla giustizia attraverso il patrocinio gratuito, anche in deroga ai limiti di reddito, e un supporto burocratico garantito da *tutor* nominati dalle prefetture. La dimensione economica, però, non è l'unica rilevante in questo disegno di legge. La nostra proposta, infatti, non vuole solo essere un atto di solidarietà, ma anche un primo passo stabile verso un approccio più strutturato e responsabile nella gestione delle infrastrutture. Promuove infatti una maggiore attenzione nella selezione delle opere pubbliche, nella loro manutenzione e nella vigilanza, chiedendo a istituzioni e operatori privati, che gestiscono beni pubblici, di assumersi pienamente la responsabilità di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Come dicevo inizialmente, infatti, il riferimento alla tragedia del ponte Morandi non deve farci dimenticare altre vicende che sono meno note, ma altrettanto gravi. Eventi simili, purtroppo, si sono verificati infatti anche in altre parti del Paese, mettendo in evidenza un problema che evidentemente non è sporadico, singolo, ma strutturale. Dunque, con questa legge vogliamo dare una risposta sistemica, riconoscendo che ogni vita persa a causa dell'incuria da parte di chi è responsabile di un'opera pubblica è inaccettabile. È una tragedia, ma è anche una sconfitta per lo Stato. Dobbiamo e vogliamo riaffermare il valore della vita umana, della dignità e della solidarietà come principi fondanti della nostra Repubblica. Ecco perché votare a favore di questa legge significa dire sì a una visione di Stato che non dimentica, che riconosce i propri errori e si impegna a fare meglio. Significa dire sì a un'Italia più sicura, più giusta e solidale. È nostro dovere morale e istituzionale garantire che le vittime non siano lasciate sole e che tragedie come quella del ponte Morandi non si ripetano più. Mi lasci ringraziare, Presidente, il ministro Salvini e nuovamente il vice ministro Rixi per aver condotto il percorso che ha portato ad un testo condiviso. Mi lasci ringraziare tutti coloro i quali, mettendo da parte ogni elemento di divisione, hanno permesso di raggiungere questo importante risultato. Un grazie anche al comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi, alla loro presidente, Egle Possetti, per non avere mai smesso di lottare per la giustizia.

credo che molti di voi abbiano in testa quei ricordi, molti si ricordano quelle emozioni forti che hanno impresso quel ricordo nella mente di ciascuno di noi. Per chi è cresciuto invece in quei quartieri, per chi è è cresciuto nel territorio genovese, per chi ha attraversato quel ponte migliaia di volte, questo è ancora più forte e indelebile nella memoria. I ricordi di quei tragici minuti sono per noi qualcosa che ci segnerà per il resto della nostra vita, noi che abbiamo la fortuna di raccontare che saremmo dovuti transitare lì quel giorno che avremmo dovuto percorrere quel ponte, ma 43 vittime innocenti e le loro famiglie non possono dire altrettanto. Non è semplicemente crollato un ponte, si sono spezzate 43 vite umane; si è sgretolato per sempre il patto di fiducia tra lo Stato e la cittadinanza, si è creata una frattura, una lacerazione profonda nella comunità. La ricostruzione del ponte ha sì ricucito la viabilità, ma non può lenire il dolore di chi ha perso una persona cara, non può restituire quelle 43 vite spezzate. Sono vittime di un drammatico intreccio di incuria, colpevoli omissioni e allarmi ignorati. Nel processo che sta portando avanti la ricerca della verità, c'è un enorme e complesso lavoro. Lo rispettiamo per l'imparzialità con cui deve essere svolto, ma in quest'Aula oggi non possiamo tacere questa vergogna nazionale, che vede alla sbarra appartenenti a società concessionarie dello Stato e a parti che appartenevano e appartengono agli uffici pubblici: un insieme di mancanze, carenze, incompetenza e delinquenza che ha permesso che quel giorno segnasse la fine per 43 persone che avevano il diritto di vivere ancora la loro esistenza. Ho voluto usare queste parole forti del Comitato dei familiari delle vittime, perché forti sono le emozioni che nascono parlando con loro: affiorano insieme rabbia, passione, amore, il ricordo dei propri cari, vittime di quella maledetta tragedia e sempre, prima di ogni altra cosa, la forte domanda di giustizia. Familiari che, riuniti nel comitato presieduto con generosità e intelligenza da Egle Possetti, svolgono un ruolo prezioso di coscienza civile, dignità, memoria e lotta, verso il quale possiamo solo esprimere gratitudine e ammirazione. Da loro nasce questa proposta di legge, a loro va riconosciuto tutto il merito. Avrebbero potuto vedere subito riconosciute a loro favore forme di sostegno, ma hanno declinato con grande determinazione e dignità; loro, che sono stati le vittime, hanno allargato lo sguardo, si sono caricati sulle spalle l'onere di ricucire quella frattura sociale, proponendo di istituire lo *status* di vittime dell'incuria come dono per il futuro, segno del lavoro fatto e dell'impegno portato avanti in questi anni. La proposta di legge che ho presentato, così come quella dei colleghi, nasce da loro, che l'hanno pensata, voluta ed elaborata partendo dal loro drammatico vissuto e da alcune misure che già oggi si applicano ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Il principio su cui tali disposizioni si fondano è quello della solidarietà sociale, sulla base del quale l'intervento dello Stato in termini di sostegno alle vittime costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica, anche in virtù della diffusa percezione che determinati eventi, sebbene colpiscano direttamente solo alcuni cittadini, a ben vedere offendono indirettamente l'intera comunità civile. Per questo abbiamo individuato una serie di misure che possono andare incontro ad alcune delle principali esigenze con cui devono confrontarsi le vittime di tali accadimenti, prevedendo forme di contribuzione economica a favore delle famiglie delle vittime, nonché la possibilità di attivare ulteriori iniziative di solidarietà sociale nei loro confronti. Per raggiungere il risultato di quest'oggi abbiamo lavorato, insieme a tutte le forze politiche, ad una proposta condivisa e credo che sia giusto, anzi doveroso, rivolgere dei ringraziamenti. Il primo al vice ministro Rixi e al ministro Salvini: ieri ho usato parole molto dure sul codice della strada, ma anch'io devo riconoscere che grazie a loro si sono messi insieme tutti e grazie a loro si è accelerato per avere un testo condiviso. Al Al presidente Balboni e alla relatrice Spinelli: anche con loro non mancano a volte motivi di scontro, ma l'umanità e la serietà istituzionale dimostrate in questa vicenda devono essere riconosciute e valorizzate.

sente la mia commozione, per essere nato e cresciuto in quel luogo, ma credo che non sia soltanto di chi è nato lì. È una tragedia che poteva e doveva essere evitata. Proprio per questo vorrei esprimere, a nome mio e dell'intero Partito Democratico, vicinanza e sostegno ai familiari delle vittime, Siamo al vostro fianco nella domanda di giustizia e confidiamo nel lavoro della magistratura per accertare pienamente ogni responsabilità su quanto accaduto. Come ha ricordato il presidente Mattarella, il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto è successo. Il 14 agosto 2018 rappresenta uno spartiacque incancellabile nella storia recente del Paese, una pagina nera per tutti e qualcosa di dolorosamente inimmaginabile per chi ha perduto qualcuno a cui voleva bene. Non possiamo cancellare il passato, ma oggi scriviamo un piccolo, piccolissimo passo per riconoscere le colpe dello Stato e impegnarlo affinché quanto accaduto non si ripeta mai più.

Signora Presidente, è inutile nascondere le emozioni che si provano oggi nel votare e nell'approvare questo provvedimento. Non è un caso che oggi la maggior parte dei senatori intervenuti siano liguri di provenienza e che il Vice Ministro oggi presente sia ligure di provenienza, non perché il fatto da cui poi è sorta la volontà di arrivare al traguardo odierno abbia interessato solo la Liguria, ma perché chiaramente i liguri sono stati colpiti. E i liguri che, come me, come il vice ministro Rixi e come gli altri rappresentanti che sono intervenuti oggi, ricoprivano già funzioni pubbliche sono stati colpiti doppiamente. Io all'epoca ero assessore ai trasporti e percorrevo quel ponte due volte al giorno, per recarmi in Regione Liguria. Il senso di vuoto, di dolore, di rabbia, di incredulità che ha colpito tutti noi quel giorno e tutti i giorni successivi

quello che stava succedendo in tutta Italia; ha messo in evidenza che le nostre infrastrutture in alcuni casi erano superate e che le infrastrutture di una Regione piccola come la Liguria sono fondamentali per il sistema economico e dei trasporti italiani ed europei, perché è ancora visibile oggi cosa è successo in tutti i giorni, i mesi e gli anni successivi fino alla realizzazione del ponte San Giorgio.

a causa dell'incuria, che finora è un concetto che giuridicamente non è mai stato utilizzato per inquadrare tragedie.

ancor prima che la giustizia, che noi speriamo arrivi presto, indichi e punisca i colpevoli che hanno causato quella tragedia. Basta dimostrare Basta dimostrare il nesso causa-effetto tra l'incuria e il disastro, e quindi le vittime susseguenti al disastro, affinché lo Stato dia un un risarcimento che, al di là dell'entità economica dello stesso, io e il Gruppo Fratelli d'Italia reputiamo importante,

L'incuria - scusate il gioco di parole che non si dovrebbe fare in questi casi - va curata; l'incuria va prevenuta con l'impegno di tutti. L'incuria non è il frutto della colpa di qualcuno, ma del disinteresse di molti. Noi oggi diciamo che il disinteresse crea una responsabilità morale dello Stato ed è un passo molto, molto importante, perché va al di sopra della sete di incolpare qualcuno, ancor prima che la giustizia abbia fatto il suo corso. Si responsabilizza il pubblico e il privato, non solo i concessionari, ma anche tutte quelle infrastrutture che sono utilizzate dallo Stato per dare servizi. Quindi tutti i servitori dello Stato, tutti coloro che amministrano il bene pubblico, devono sapere che la loro incuria, il loro disinteresse, sebbene non sia un reato (perché l'incuria non è reato), ha come conseguenza un danno per lo Stato e questo, oltre al danno morale di creare vittime e quindi di perdere cittadini, prevede un risarcimento e quindi comporta un costo. Dobbiamo evitare per prima cosa che ci siano ulteriori disastri. Dobbiamo garantire la sicurezza dei cittadini; dobbiamo garantire che lo Stato

di silenzio assordante che abbiamo provato noi liguri il 14 e il 15 agosto del 2018 e tutti i giorni, le settimane, i mesi e gli anni successivi. Sono sensazioni che si provano ancora adesso tutti gli anni il 14 agosto, quando andiamo sotto l'attuale ponte San Giorgio a ricordare quello che è successo. La memoria di quanto è accaduto, infatti, è alla base del provvedimento che oggi noi andiamo a votare, ma anche della responsabilizzazione che tutti noi che facciamo politica e amministriamo il bene pubblico dobbiamo avere e dobbiamo trasmettere alle future generazioni. Anche io desidero ringraziare tutti i Gruppi parlamentari che hanno voluto, in un solo provvedimento, significare la volontà della politica di fare qualcosa al di là

nn. 794 e 868, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale».

tutta l'Assemblea, la relatrice, il presidente Balboni, il Vice Ministro e il Governo perché, nonostante non ci sia alcun risarcimento che possa ripagare le 43 vittime, questo è un atto di giustizia, come hanno ricordato tanti colleghi, perché non accada mai più quello che è accaduto quel 14 agosto. Grazie veramente a tutti.

senatrice Malpezzi, la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione è prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La garanzia di tale servizio a favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, spetta ai Comuni. In Lombardia i Comuni costituiscono con risorse proprie, anche per assicurare il servizio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'istruzione e formazione professionale, su deroga della Regione, come previsto dalla legge regionale n. 31 del 26 maggio 2017. Tanto premesso, l'ufficio scolastico regionale della Lombardia ha evidenziato che, riguardo alla difformità tra la richiesta di ore di assistenza previste nel piano educativo individualizzato (PEI) e le ore effettivamente riconosciute dall'ente locale, sono intervenute numerose sentenze di segno non univoco dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato. In effetti, mentre per il sostegno didattico la giurisprudenza è unanime nel ritenere che non è accettabile un vincolo derivante dalla carenza di risorse finanziarie, non sempre ciò è stabilito nel caso dei ricorsi delle famiglie degli studenti con disabilità, ai quali i Comuni, per ragioni finanziarie, non garantiscono l'intero servizio di assistenza richiesto nel PEI. Particolarmente significativa è la sentenza del Consiglio di Stato n. 7089 del 12 agosto scorso, secondo cui il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è da intendersi come un servizio di supporto per il quale gli enti locali potrebbero potrebbero assegnare le ore nei limiti delle risorse disponibili, diversamente dal sostegno didattico, che invece rientra nell'ambito del diritto allo studio e all'istruzione, al quale la Costituzione garantisce un valore fondamentale. In questo quadro complesso e in via di trasformazione, è chiaro che le problematiche relative alla garanzia di tale servizio non riguardino solo il Comune di Sesto San Giovanni, ma rappresentino piuttosto una questione generale relativa a tutto il sistema delle autonomie locali, come peraltro si evince chiaramente, se ci limitiamo alle specificità della Lombardia, dalle iniziative svolte dalla locale componente di ANCI. Chiarito ciò e chiarito che la competenza è degli enti locali, voglio segnalare che questo Governo sta facendo anche in questo ambito il suo dovere, proprio per affrontare un tema di cui riconosciamo l'importanza fondamentale. Proprio in questi giorni, infatti, sta entrando nel vivo l'esame presso la 7a Commissione di questo ramo del Parlamento di più proposte di legge parlamentare sostenute dal Governo, il cui obiettivo è quello di colmare le lacune originate dalla mancata attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che avrebbe dovuto, tra le altre cose, disciplinare la rinnovata figura dell'assistente alla comunicazione. Prendendo atto del fallimento di quella riforma, il Governo è ora al lavoro insieme alle forze parlamentari per individuare il giusto livello di formazione e di retribuzione per queste figure insostituibili per il benessere dei nostri studenti con disabilità. A prescindere dai prossimi interventi riformatori della materia, aggiungo che nel frattempo il Ministero ha comunque rafforzato le proprie azioni rispetto al passato, al fine di assicurare il diritto allo studio dello studente con disabilità. La principale competenza del Ministero in questo ambito è infatti quella di reclutare e formare docenti specializzati sul sostegno in grado di promuovere il pieno processo di inclusione degli studenti con disabilità. Ebbene, desidero ricordare che per garantire tale diritto il Ministero ha, in questi due anni, svolto azioni eccezionali. Mi riferisco, in particolare, alla procedura speciale per le immissioni in ruolo riservata ai docenti inseriti nella prima fascia da GPS su posto di sostegno per l'anno scolastico 2023-2024, che ha fatto registrare una percentuale pari al 74,1 per di copertura dei posti di contingente sul posto di sostegno rispetto al 53,2 per cento di copertura nell'anno scolastico 2022-2023, per un totale di circa 18.000 posti autorizzati su sostegno. Tale procedura è stata peraltro ripetuta anche per questo anno scolastico, pure in concomitanza con l'avvio delle nuove procedure di reclutamento previste dal PNRR e ha favorito l'assunzione di docenti di sostegno proprio nelle Regioni del Nord, dove i concorsi non avevano raggiunto la copertura dei posti messi a bando per assenza di candidati. Concludo che, sempre al fine di assicurare il supporto di docenti sempre più qualificati, il Governo è intervenuto in modo estremamente significativo e concreto, agendo alla radice delle cause che non hanno consentito in tutti questi anni che vi fosse un sufficiente numero di docenti specializzati sul sostegno, soprattutto al Nord. Si deve infatti a questo Governo la scelta di introdurre un nuovo sistema di specializzazione sul sostegno rivolto a chi già da anni assicura questo servizio, per quanto in modo precario. A questi docenti, finalmente, è stata data la possibilità di qualificarsi ulteriormente e di conseguire la specializzazione, in modo da poter partecipare ai concorsi che, come detto, conoscono gravissime carenze di candidati proprio nelle Regioni del Nord e in particolare in Lombardia.

che, come in tante altre realtà d'Italia - in questo caso a Sesto San Giovanni, ma potremmo citarne altre - riguarda delle famiglie che si trovano ad avere dei figli disabili a cui, nel piano educativo individualizzato, vengono riconosciute una serie di ore sia per il sostegno, sia per l'assistenza alla comunicazione e ai quali poi queste ore non vengono date. A quel punto a quelle famiglie,

cause legali contro il Ministero. Siccome sono una donna delle istituzioni, sono sempre preoccupata quando queste diventano oggetto di cause

Al netto di tutto questo che è brutto - dobbiamo dircelo che è brutto, perché vuol dire che ci sono dei genitori che per vedere il diritto garantito ai loro figli fanno causa a un Governo o, meglio, a uno Stato che dovrebbe tutelarli e quindi, chiaramente, io mi scaldo per questo

dovremmo rispondere non nel modo in cui ha risposto lei. Lei ha affermato che il Consiglio di Stato ha detto che alla fine alle ore di autonomia devono pensare i Comuni e non lo Stato. Bene, i Comuni con che soldi affrontano il discorso dell'autonomia educativa ai ragazzi? Se tagliamo i trasferimenti ai Comuni e se poi magari in un Comune in quelle annate il numero dei ragazzi con disabilità è più alto, questi Comuni come caspita riescono a fare il bilancio? Avremmo dovuto prendere la sentenza - perché le sentenze non si commentano, una volta che ce l'hai, la prendi - e avremmo dovuto dire tutti insieme che dobbiamo fare in modo che l'autonomia educativa venga garantita, aumentiamo i trasferimenti ai Comuni, cerchiamo di fare in modo di capire con quale modalità possiamo sostenerli per consentire a quelle famiglie e, quindi, a quei bambini di avere il loro diritto all'istruzione garantito dalla Costituzione, di cui tutti noi dovremmo essere custodi. La prima risposta che mi sarei aspettata è questa: lavoriamo insieme per maggiori trasferimenti. Il problema è che anche a questo giro nella di bilancio i trasferimenti agli enti locali vengono tagliati e non aumentati. Questa è però un'altra storia e ci saranno altri ambiti su cui intervenire. Aggiungo però un altro elemento. Capisco tutta la difficoltà del mondo del sostegno e dico, con altrettanta onestà intellettuale, che non inizia con il Governo di Giorgia Meloni perché quel problema è annoso, lo abbiamo da sempre. Il numero degli insegnanti di sostegno è infatti minore di quanto sia la necessità e il bisogno. Possiamo anche dirci però che poter diventare insegnanti di sostegno costa tantissimo e che le università non aprono tutti i corsi e i percorsi per poter fare in modo di ottenere questo tipo di formazione? Noi, che abbiamo bisogno di insegnanti di sostegno, gli diciamo di specializzarsi, pagando però 2.500 euro. Vi sembra una cosa normale? Questo sistema non funziona più. Allora o diciamo che prendiamo in mano la nostra legge molto innovativa - nostra nel senso di Parlamento italiano - sull'inclusione scolastica e ricordiamo sempre che il sostegno è un sostegno alla classe e che quindi noi dovremmo fare in modo di potenziare tutti gli insegnanti,

che la classe sia davvero inclusiva e rispetteremo davvero la volontà di quella legge che ha fatto scuola in tutta Europa, ma che purtroppo rimane ancora incompiuta.

finestra") sulle condizioni detentive delle carceri italiane, in particolare nel penitenziario di Regina Coeli di Roma. Signor Presidente, senatrice D'Elia, l'atto di sindacato ispettivo solleva specifici quesiti in ordine ad asseriti aspetti di criticità della casa circondariale di Roma Regina Coeli, con particolare riguardo alle carenze degli organici e al tasso di affollamento della struttura. L'attenzione al sistema carcerario è tra le priorità di questo Dicastero e del Governo. È nostro dovere perseguire un modello di carcere che assicuri un'esecuzione della pena certa e, al contempo, mai lesiva della dignità umana; un modello di carcere vivibile sia per chi vi è recluso, sia per chi ci lavora. Come ha più volte ribadito il ministro Nordio la linea di questo Governo è puntare sull'umanizzazione della pena. Queste due direttrici hanno orientato l'azione del Governo Meloni, che con il decreto-legge 4 luglio 2024, 2024, n. 92, cosiddetto carcere sicuro, ha dato risposte straordinarie ed energiche all'emergenza del sovraffollamento, ma anche soluzioni adeguate, proporzionali e lungimiranti ai problemi strutturali, trascinati da anni dal sistema penitenziario. Per quanto riguarda le carenze di organico della casa circondariale di Regina Coeli, le notizie acquisite presso il DAP riferiscono che, a fronte di un organico previsto di 480 unità, la forza presente è pari, allo stato, a 350 unità, inferiore dunque rispetto a quella prevista di complessive 130 unità. In particolare, le carenze di organico della Polizia penitenziaria si rilevano nel ruolo dei funzionari (meno una unità), nel ruolo degli ispettori (meno sei unità), nel ruolo dei sovrintendenti (meno tre unità); di contro, il ruolo degli agenti assistenti risulta in esubero di un'unità. Dall'insediamento di questo Governo la casa circondariale di Regina Coeli ha avuto un potenziamento dell'organico. In particolare, nel ruolo agenti assistenti sono state inviate 24 unità dalla mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni del 181° corso; 3 unità dalla mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni del 182° corso; 19 unità dalla mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni del 183° corso. A gennaio 2025 saranno assegnate ulteriori 1.713 unità del 184° corso e le esigenze dell'istituto di Regina Coeli saranno debitamente tenute in considerazione dall'amministrazione. La casa circondariale di Regina Coeli è retta da un direttore, due vicedirettori e da un comandante titolare, una situazione che rafforza significativamente la catena di comando e che è di fondamentale importanza nella gestione di un istituto penitenziario delicato come questo. Con le nuove assegnazioni di dirigenti penitenziari è previsto l'invio di un terzo vicedirettore. Per quanto riguarda l'area trattamentale, si segnala che la pianta organica relativa ai funzionari giuridico-pedagogici risulta pienamente soddisfatta, con 11 presenze effettive su una previsione organica di 11 unità. Sin dal suo insediamento il Governo Meloni ha adottato una serie di interventi volti a potenziare l'organico e le dotazioni della Polizia penitenziaria del comparto funzioni centrali. Per quanto riguarda il Corpo della Polizia penitenziaria segnalo sinteticamente alcuni degli interventi più significativi che sono approntati. Per quanto riguarda il ruolo dei commissari del Corpo, vi è il concorso per 120 posti, attualmente in formazione, che saranno inviati, e l'assunzione di ulteriori 22 unità tramite scorrimento della

che saranno assegnati alle sedi a maggio 2025, e l'assunzione di ulteriori 48 unità tramite scorrimento della graduatoria, come previsto dal decreto-legge n. 92 del 2024. Per quanto riguarda il ruolo degli agenti assistenti, sono state assunte 1.479 unità del 181° corso, assegnate nel luglio 2023; 244 unità del 182° corso, assunte mediante lo scorrimento delle graduatorie e assegnate ad aprile 2024; 1.870 unità del 183° corso, assegnate l'8 luglio 2024; 1.713 unità del 184° corso, che stanno terminando il corso di formazione e saranno assegnate entro febbraio 2025; un concorso per nuovi 2.568 allievi

concorso per 52 dirigenti penitenziari, che prenderanno servizio nelle sedi a dicembre 2025; un ulteriore scorrimento della graduatoria per 12 unità, avviate al corso di formazione di consigliere che ha avuto inizio l'8 luglio 2024. Grazie a queste assegnazioni sarà possibile garantire un direttore titolare per ogni istituto e, negli istituti più complessi, anche la presenza in pianta stabile del vicedirettore. Significativo è anche lo sforzo assunzionale del comparto funzioni centrali, concorso per 104 funzionari giuridico-pedagogici, il concorso per 140 funzionari contabili, i cui vincitori hanno preso servizio il 16 gennaio 2023, un ulteriore concorso per 107 funzionari contabili; dei 135 idonei purtroppo solo 77 hanno accettato la sede e sono stati assunti in servizio dal 29 luglio 2024. In data 24 ottobre 2024 è stato bandito un concorso per ulteriori 77 unità; concorso per 37 funzionari tecnici, che prenderanno servizio a dicembre 2024, andando a saturare la pianta organica di tale famiglia; assunzione di 58 unità, su una pianta organica di 67, per funzionari di mediazione culturale. un primo concorso per 203 assistenti tecnici e un secondo concorso per ulteriori 150 unità, attualmente in svolgimento; per i contabili di Area II, assunzione di 45 unità e, attualmente in svolgimento, un concorso per altre 50 unità; per gli assistenti amministrativi, l'assunzione di 12 unità a scorrimento e graduatoria per ulteriori 80 unità, attualmente in fase di assegnazione delle sedi. Anche di queste misure si potrà presto giovare la casa circondariale di Roma Regina Coeli. Per quanto riguarda, invece, le presenze detentive presso la casa circondariale Regina Coeli, alla data del 14 novembre 2024 sono presenti un totale di 1.124 detenuti a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi 628 posti disponibili, con un indice di affollamento pari al 198,59 per cento, che purtroppo costituisce la percentuale più alta dell'intero distretto. Nonostante il dato rappresentato, non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte EDU, in quanto i detenuti si trovano in spazi compresi tra i 3 e i 4 metri quadrati. Ad ogni buon conto, al fine di alleggerire la pressione detentiva sulla popolazione carceraria presente, sono stati recentemente adottati, dalla Direzione generale dei detenuti del trattamento, provvedimenti deflattivi che hanno portato a trasferimenti di detenuti dalla casa di Regina Coeli verso istituti penitenziari di Viterbo, Chieti, Frosinone, Cassino e Pescara. Per quel che concerne l'offerta trattamentale dell'analisi del progetto pedagogico relativo all'anno si rileva che nell'istituto sono attive numerose iniziative formative, sia di istruzione sia di corsi professionali, nonché numerosi progetti e laboratori dedicati ad attività teatrali, artistiche e musicali. Quanto, infine, al triste dato dei suicidi dall'inizio del 2020 ad oggi, presso l'istituto di Roma Regina Coeli si sono purtroppo verificati 13 suicidi tra la popolazione detenuta. Come più volte ribadito, il tema della prevenzione del suicidio costituisce un persistente punto di interesse, fulcro di attività da parte del Ministero, che si è impegnato a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi e di misure in questo ambito. Al riguardo, è attivo un percorso nazionale di intervento continuo sul tema, attraverso il quale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi sono coinvolti in una prospettiva di rete nella prevenzione di tali drammatici Su questa linea assume un ruolo fondamentale lo *staff* multidisciplinare, al punto di essere stato istituito uno specifico gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi degli eventi suicidari delle persone detenute, con il compito di definire protocolli operativi ed elaborare momenti di formazione per il personale penitenziario, al fine di tutelare la salute psicofisica dei detenuti e prevenire i suicidi. Signor Presidente, signor Sottosegretario, qui davvero non ci siamo. Modello di carcere vivibile, risposta straordinaria, lungimiranti?

Mai, come nel caso delle carceri, i numeri sono persone e spazi di vita che, in un universo concentrazionario quale quello carcerario, sono la vita. Tutto quello che avviene dentro quelle mura conosce da sempre la tirannia del dato, la sua implacabile durezza, prima degli algoritmi e delle schiavitù digitali. Abbiamo riportato dei Abbiamo riportato dei numeri nella nostra interrogazione. Lo ha fatto la senatrice D'Elia, che ringrazio per il tempo di parola affidatomi. Credetemi, è cosa rara in politica questa generosità. Tali numeri non lasciano grandi margini di giustificazione a questo Governo. I concorsi, lo scorrimento delle graduatorie, le assegnazioni: ma di cosa stiamo parlando? presentammo il nostro atto, signor Presidente, i detenuti nelle carceri italiane erano 61.049, secondo i dati di Antigone, a fronte di una capienza ufficiale stimata in 51.178 posti. A ottobre sono diventati 62.110. Siamo al 132,3 per cento rispetto alla capienza regolamentare disponibile. Quando, insieme ai parlamentari Caso e Madia, andammo a fare visita al carcere di Regina Coeli, il tasso di sovraffollamento sfiorava il 182 per cento. Oggi quella stessa cifra è salita, come ha detto adesso il Sottosegretario, al 198 di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale. Cosa è successo in questi mesi? Un inutile decreto sulle carceri da parte del Governo, una faccia feroce, priva di qualsiasi apprezzabile conseguenza per i cittadini, ma che purtroppo ha avuto un ulteriore impatto negativo, un incrudelimento sulle condizioni di vita dei detenuti. Questa notte, Presidente, a Poggioreale si è tolto l'ottantunesimo detenuto dall'inizio dell'anno. Si è impiccato, si è tolto l'aria, l'ossigeno! A questi vanno sommati sette operatori carcerari che si sono suicidati in questo anno. Sono stati 1.842, a oggi, i tentativi di suicidio e 11.503 gli atti di autolesionismo. Una guerra. Le carceri si riempiono e soffocano - la mancanza d'aria orgogliosamente rivendicata dalle ignobili parole del sottosegretario Delmastro - di persone che spesso, semplicemente, non dovrebbero stare lì. Quindi pattuglioni che sbattono in galera un po' di gente non danno una risposta, una, efficace, utile, efficiente e apprezzabile alla richiesta di sicurezza che viene dalle persone. Sono più sicuri oggi gli italiani? No, Presidente. Sono

di clemenza. Stefano Anastasìa, il Garante dei detenuti del Lazio, ha chiesto di sospendere gli ingressi negli istituti più congestionati come il carcere romano. In questi mesi ci sono state crescenti tensioni a Regina Coeli: una trappola di metallo - vi inviterei a visitarla - che sta alla dignità della detenzione come il sottosegretario Delmastro sta alla dignità dell'istituzione che, speriamo ancora per poco, rappresenta. E non andare via, Roberto, non andare via. *(**Applausi*.*Commenti)*. Risse, scontri, incendi, danni; è stata chiusa la famigerata ottava sezione. Sono episodi che segnalano la criminalità di chi è detenuto, ma l'inumanità in cui scontano la loro pena i detenuti e le difficoltà estreme in cui si trova a operare il personale carcerario. Siamo in un concentrato foucaultiano invivibile per i detenuti e gli operatori e gli operatori sotto-organico. La Polizia, alla quale digrignate sempre la vostra vicinanza, non potrebbe essere lasciata più sola e abbandonata su quella frontiera. Colleghi, quello che avviene nelle carceri non misura soltanto il livello di civiltà, democrazia e libertà di una Nazione (la Nazione, come amate dire voi), ma sta in un equilibrio da vasi comunicanti con chi sta fuori. Non è filosofia, ma fisica. Per quanto alti siano i muri e remote e inaccessibili le carceri, le condizioni di chi è là dentro non solo ci riguardano, ma affettano la vita di tutta la comunità. Non pensate di chiudere fuori il rifiuto, lo scarto, l'osceno. E non solo perché sono persone e cittadini, ancorché alcuni non abbiano la cittadinanza italiana, insistono e vivono nelle nostre città, con buona pace di tutte le Albanie del mondo, e continueranno a farlo. Quello che succede nelle nostre carceri si scarica sulla vita quotidiana di chi sta fuori. Carceri non sicure significano una società meno sicura; carceri senza diritti significano una società con meno diritti, dove è più facile perderli o non accorgersi che li stiamo perdendo. È paradossale che una lezione sulla nostra libertà ci venga da chi è ristretto, da chi ha perso la propria libertà e la agisce con limitazioni fisiche. Concludo. Non è filosofia o sociologia, è fisica meccanica dei corpi, dinamica dei fluidi, ragion per cui queste queste vostre misure (e anche la sua risposta, Sottosegretaria) non rispondono alla richiesta di sicurezza dei cittadini e degli italiani, proprio perché rendono meno degne, civili e sicure le nostre carceri e, dunque, la nostra società, le nostre città, le nostre vite. *(Applausi)*.

con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante chiede chiarimenti in merito all'ipotesi di una cessione della struttura della casa circondariale di Lanusei, attualmente rientrante nel patrimonio immobiliare del DAP, al Dipartimento per la giustizia minorile di comunità, perché possa utilizzarsi come struttura per detenuti minorenni. A corredo di tali ipotesi, l'interrogante associa anche l'ulteriore circostanza che sarebbe stata individuata anche in un gruppo di detenuti minorenni, definiti piuttosto facinorosi e ribelli, da avviare alla citata struttura penitenziaria. Per quanto riguarda il delicato e complesso sistema detentivo minorile, occorre premettere che questo Governo è ben consapevole che, nei confronti della popolazione detenuta minorenne, è necessario un più attento bilanciamento tra la necessità di rendere effettiva e certa la pena e l'esigenza di una più spiccata vocazione rieducativa nei confronti dei minori ristretti. Anche in questo specifico settore, il Governo sente come priorità l'esigenza di elevare gli *standard* operativi e qualitativi della giustizia minorile, con interventi concreti a lungo termine. Occorre infatti rivisitare le misure organizzative, operative e strutturali di sicurezza degli istituti penali per i minorenni, al fine di favorire contesti formativi e di prevenire e gestire conflittualità ed episodi di violenza. Occorre premettere che anche il comparto carcerario minorile soffre una condizione di sovraffollamento, anche in conseguenza dell'afflusso esponenziale in Italia di minori stranieri non accompagnati, che quando delinquono si riversano giocoforza nel circuito penale minorile. A fronte di una capienza totale di 534, posti sono attualmente ristretti 568 detenuti minorenni, di cui 536 maschi e 32 femmine. Quasi la metà dei detenuti degli istituti penali si tratta spesso di ragazzi assuntori di sostanze stupefacenti o psicofarmaci con gravi problematiche comportamentali che finiscono per essere immessi nel circuito carcerario, anziché in apposite comunità educative ad alta intensità sociosanitaria. Proprio per dare una risposta a questa specifica critica, il cosiddetto decreto carceri del 4 luglio 2024, n. 92, ha previsto l'istituzione di specifici corsi di comunità dedicati ai detenuti degli IPM. In particolare, sono in fase di realizzazione almeno sette nuove comunità ad alta integrazione sociosanitaria, distribuite sul territorio nazionale (in particolare tre Milano, due a Roma, una Caserta e una Cagliari), per accogliere i minori con comprovato disagio psichico e dipendenze. Per due strutture in Lombardia sono state concluse le gare d'appalto, mentre per le altre sono in fase di avvio le procedure previste. Mi permetta anche di sottolineare che alcune criticità sono ampiamente imputabili alle conseguenze derivanti dalle decisioni politiche adottate dai precedenti Governi, come quella di mantenere nelle strutture detentive minorili i condannati fino al compimento del venticinquesimo anno di età, circostanza che mette in pericolo il percorso rieducativo della popolazione detenuta più giovane, surrogata dalla negativa influenza criminale dei ristretti più adulti. Per affrontare questo fenomeno, ad esempio, nell'ambito del cosiddetto decreto Caivano, il Governo ha adottato opportune misure che permettono, previa valutazione personalizzata del magistrato, il trasferimento per adulti di quei detenuti maggiori di ventuno-diciotto anni che si macchiano delle seguenti condotte: tenere comportamenti che compromettono la sicurezza o turbano l'ordine degli istituti; fare uso di violenza o minaccia per impedire le attività di altri detenuti; avvalersi dello stato di soggezione generato degli altri detenuti. Venendo nello specifico dei quesiti riportati nell'atto di sindacato ispettivo, colgo l'occasione per informare con chiarezza e certezza che è tassativamente esclusa ogni ipotesi di trasferimento, sia essa anche solo temporanea, di un contingente di detenuti minorenni presso le strutture della casa circondariale San Daniele di Lanusei, che rimarrà dunque casa circondariale destinata alla popolazione adulta. Dai contributi forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è emerso che il suddetto istituto è stato oggetto di attenta valutazione di idoneità da parte di un'apposita commissione, costituita il 7 giugno 2024, dal direttore generale del personale del Dipartimento di giustizia minorile. L'attività di ricognizione svolta per stabilire se la casa circondariale di Lanusei potesse essere destinata a istituto penale per i minorenni ha avuto dunque esito negativo. Tale ipotesi è stata definitivamente scartata, tanto che, esaminando la relazione di sopralluogo, svolto il 10 giugno 2024 dalla direzione

tra cui la casa circondariale di Lanusei, per contingenti esigenze legate alla dismissione, nel passato, di importanti compendi detentivi minorili all'avvio, e nel presente, della ristrutturazione di ben cinque istituti penali minorili e alla cronica insufficienza di comunità socioeducative sul territorio nazionale. Con nota del 30 luglio 2024 il Dipartimento di giustizia minorile ha poi ritirato la succitata richiesta, comunicando che, in esito a preliminari verifiche conoscitive, ha potuto accertare l'assoluta incompatibilità del carcere San Daniele di Lanusei con la destinazione della medesima struttura a IPM DGMC e pertanto dismette l'ipotesi avanzata. Confermo quindi che la predetta struttura penitenziaria rimarrà in uso all'amministrazione penitenziaria quale casa circondariale di Lanusei.

sottosegretaria, la ringrazio per la risposta, per le informazioni e per le rassicurazioni, che fanno seguito, tra l'altro, a un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera, che chiedeva al chiedeva al Governo di scongiurare il trasferimento, anzi la deportazione di un numero di ragazzi detenuti a Lanusei. Ne prendo atto, ma noi non ci fidiamo, perché lei stessa ha confermato come questa ipotesi fosse stata perseguita: c'erano stati un sopralluogo e una valutazione. Non voglio esagerare nei termini, ma la stampa sarda, che ha denunciato (questo è il termine giusto) questa ipotesi, aveva parlato, senza esagerare troppo, di Guantanamo, perché la vostra logica è quella. Lei ha parlato delle carceri minorili di questo Paese descrivendo queste situazioni in maniera quasi asettica. Ma lei non può non sapere che, soprattutto con le vostre scelte, con l'aumento e la definizione di nuovi reati,

se ieri abbiamo avuto la notizia che cinque concorsi per direttori di istituti minorili sono andati deserti. È evidente che, se riempite le carceri minorili di ragazzi ai quali viene negata in quelle sedi ogni possibilità di istruzione così come gli è stata negata in gran parte nella loro vita quotidiana, se non combattete la dispersione scolastica e se non offrite loro occasioni di lavoro e di vita sociale definita soprattutto in certe zone, credo

il suo debito con la giustizia (come è giusto che avvenga), ricordatevi che l'articolo 27 della Costituzione e soprattutto i principi di umanità impongono di di stabilire una pena che abbia fini rieducativi e riabilitativi, non di vendetta, non di afflizione, non di gusto sadico, come abbiamo letto nelle vergognose, deliranti, ma purtroppo consapevoli parole del sottosegretario Delmastro che aveva quasi il gusto di non far respirare dei detenuti macchiatisi di qualche reato. *(Applausi)*. Non ci stanchiamo di ripeterlo: con con queste politiche di vendetta e non di recupero voi minate anche la sicurezza dei cittadini, perché un detenuto che ha sbagliato, che paga il suo debito e che esce rieducato non torna a delinquere. Invece, nel momento in cui tenete le prigioni in questo stato di sovraffollamento e in queste condizioni (stamattina

come ha scritto benissimo oggi Lirio Abbate su «la Repubblica», sappiamo anche per esperienza diretta che la stragrande maggioranza degli agenti di Polizia penitenziaria va solo ringraziata per il lavoro difficile che fa. Ma la teoria delle mele marce rischia di non bastare più, perché le mele - come ha scritto Lirio Abbate oggi - marciscono se l'aria in cui si trovano è cattiva; e se l'aria è quella praticata, diffusa predicata dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove, le mele marciscono sempre di più. Voglio davvero chiudere, signor Presidente, e mi scuso se ho preso un minuto in più. Oggi c'è stato un altro bellissimo intervento di una persona che ha speso la vita fondando Antigone, l'associazione che che si occupa del lavoro dentro le carceri; mi riferisco a Patrizio Gonnella, il quale, in un articolo su «il manifesto», ha scritto una cosa davvero importante. Egli dice

in tutta Italia, sono costantemente effettuate dalle Forze dell'ordine. La tematica è affrontata sistematicamente nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica, ove sono state delineate le seguenti linee di intervento volte a rafforzare l'attività l'intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio con la presenza di personale del reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato per periodi prolungati; l'utilizzo di aliquote di Compagnia di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri; lo svolgimento di operazioni ad alto impatto con controlli capillari e mirati nelle zone ritenute maggiormente a rischio; la comunicazione alla cittadinanza mediante *media* locale dell'importanza di fornire tempestiva segnalazione di eventuali situazioni sospette alle Forze di polizia. In particolare, la Polizia di Stato, oltre all'ordinaria attività, ha svolto nel corso dell'anno complessivamente 84 servizi straordinari di controllo del territorio, anche con il supporto aggiuntivo degli equipaggi del reparto prevenzione crimine. I suddetti servizi sono stati estesi anche ai Comuni limitrofi a Campobasso e a Termoli, in particolare a quello di Campomarino. Quale segnale di vicinanza alle comunità locali e alle esigenze delle specifiche realtà della Provincia, la prefettura ha programmato il prossimo svolgimento di sedute del predetto Comitato decentrate sul territorio e aperte alla partecipazione dei sindaci interessati. Un'ulteriore recente iniziativa in chiave di prevenzione è costituita dal protocollo di intesa sottoscritto con Confcommercio e Confesercenti in materia di videoallarme antirapina. Preme anche sottolineare che lo scorso 30 ottobre, alla presenza del Ministro dell'interno, è stato sottoscritto un protocollo di intesa dal prefetto di Campobasso e dal Presidente della Regione, con l'adesione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Campobasso, distrettuale antimafia, e della procuratrice presso il tribunale di Larino, per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza su tutto il territorio della Provincia. Sotto il profilo attuativo, il predetto protocollo prevede l'impegno della prefettura di acquisire l'impianto di videosorveglianza e le necessarie infrastrutture, mentre la Regione Molise si è impegnata a effettuare l'attività di stazione appaltante e provvedere, con risorse proprie, alla manutenzione e alla copertura dei costi del finanziamento del sistema. Il protocollo in questione prevede inoltre l'installazione di telecamere con il sistema di lettura targhe lungo le principali arterie stradali che collegano importanti centri abitati della provincia. Tale iniziativa si salda con un'attività di controllo del territorio operata dalle Forze dell'ordine quale ulteriore fattore di deterrenza per le attività criminose. L'intensificazione delle attività di controllo del territorio coordinate dalla prefettura, unitamente alle operazioni disposte all'autorità giudiziaria, ha portato a tangibili risultati sotto il profilo del contrasto dei reati predatori. Dai dati in possesso della Polizia di Stato rilevati dall'inizio di questo anno alla data del 30 settembre 2024, nella provincia di Campobasso si registra una generale diminuzione dei furti di circa l'11 per cento rispetto all'analogo periodo del 2023, mentre nella città capoluogo il decremento si attesta intorno al 27 per cento circa. Infine si fa presente che, in relazione agli organici della Polizia di Stato, tra dicembre di quest'anno e gennaio del prossimo anno, a conclusione del 227° corso allievi agenti e del 17° corso allievi vice ispettori, verrà realizzato un piano di mobilità del personale che riguarda tutta Italia, ma che in particolare per la questura di Campobasso si articola in un incremento di dieci unità, di cui cinque del ruolo degli agenti assistenti; saranno inoltre destinati alla questura un ispettore dell'articolazione periferica del un ispettore della polizia stradale e tre unità presso la Scuola allievi agenti di Campobasso. Permangono quindi costanti l'impegno e l'attenzione della prefettura e delle Forze dell'ordine, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini mediante strategie operative volte all'intensificazione del controllo del territorio e alla prevenzione di attività criminose, che passa da una stretta sinergia con gli enti territoriali. [DELLA

io sono soddisfatto della sua risposta che mette in luce due punti. Il primo è l'attenzione del Governo alle periferie e comunque in generale al territorio dello Stato: in questo caso mi riferisco al mio Molise. Lo dico anche da sindaco di un Comune che è alle porte di Termoli, cioè San Giacomo degli Schiavoni, che è molto vicino a Campomarino, due Comuni citati nella risposta. Non posso però non ringraziare in modo altrettanto puntuale tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno difendono la nostra sicurezza in tutte le parti d'Italia. *(Applausi)*. A loro va il nostro ringraziamento.

ho ritenuto di dover intensificare gli sforzi verso un ulteriore invio di contingente militare e della Polizia di Stato. Per questo dico che la risposta del Sottosegretario delle quali attiene al protocollo d'intesa che il ministro Piantedosi ha firmato a Campobasso con la prefettura e con la Regione, per dotare tutte le arterie viarie di videosorveglianza attiva con lettura delle targhe. Ciò consentirà, ovviamente, di avere un controllo e fungerà anche da deterrente per la commissione in questo caso di reati predatori, nella fattispecie furti: furti davvero a raffica e organizzati, che non possono essere opera di un singolo. riguarda l'aumento del contingente della Polizia di Stato; un aumento anche numerico che spero nei prossimi mesi, con i nuovi concorsi, possa portare, oltre alla Polizia di Stato, anche l'aumento dei

seppur per le vie brevi, al ministro Piantedosi: quella cioè che Campobasso torni ad essere una questura di fascia A, con una dirigenza generale, perché oggi sconta il fatto di essere l'unico capoluogo di Regione che non è ancora una questura di tale fascia. Signor Sottosegretario, rivolgo quindi anche a lei questo invito e spero che possano essere al più presto accontentati non solo io, ma la Regione Molise e in particolare la città di Campobasso

dichiaro assolutamente soddisfatto della sua risposta.

la cultura*. Gentili senatori, si rappresenta che la Certosa di San Lorenzo di Padula garantisce un'ampia apertura giornaliera dalle ore 9 alle ore 19,30, più estesa rispetto alla media delle aperture giornaliere dei siti museali statali. Come nella quasi totalità dei musei del Ministero della cultura, è previsto un giorno di chiusura, che nello specifico è individuato nel martedì, sia in considerazione delle necessità connesse alle turnazioni di personale, sia per consentire lo svolgimento senza la presenza di pubblico di attività indifferibili quali manutenzione ordinaria e straordinaria e di quelle connesse con lo svolgimento dei lavori dei cantieri in corso. Rispetto alla notizia relativa ai tre pullman giunti alla Certosa nel giorno di chiusura, si segnala che gli orari di apertura, sempre aggiornati, sono comunicati al pubblico e agli operatori turistici attraverso diversi canali ufficiali di comunicazione, quali l'*app* Musei Italiani e il sito del Ministero, alla sezione dedicata ai luoghi della cultura, oltre che nella pagina di acquisto *online* dei biglietti di ingresso. Al riguardo, si rappresenta che l'*app* Musei Italiani, disponibile negli *store* già da luglio 2023, è stata pensata come utile strumento per l'organizzazione delle visite presso i luoghi della cultura del sistema museale nazionale.

sulla base di un'attenta valutazione sui flussi turistici. Tuttavia, in base alle previsioni legate alla diversa affluenza durante il corso dell'anno, sarà cura sarà cura della Direzione regionale Musei nazionali Campania individuare un giorno diverso per garantire la massima fruizione del sito. Per quanto riguarda la prospettata e auspicata apertura della sede tutti i giorni della settimana, la Direzione regionale Musei nazionali Campania ha avviato un intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza da remoto che, consentendo l'abolizione del turno notturno, permetterà di recuperare unità di personale di vigilanza e, di conseguenza, di ampliare l'offerta di fruizione del sito.

alla possibilità non solo di implementare l'orario di apertura, ma soprattutto di considerare, attraverso investimenti del Ministero, la possibilità di apertura tutti i giorni della settimana.

degli investimenti. Le spese finali per il Ministero della cultura ammontano a 3,5 miliardi, pari allo 0,4 per cento della spesa finale della finanziaria, con una riduzione di 124,2 milioni rispetto all'anno precedente.

l'economia del luogo si basa molto sulla cultura. Voglio ricordare al Sottosegretario che lo scorso 30 ottobre si è tenuto, presso la Certosa, la presentazione del modello Culturitalia, Culturitalia, un'idea da cui è nato l'articolo 31 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, volta a promuovere l'Italia o parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica. turistica. Sulla scorta di questa vostra scelta, si dovrebbe pensare di fare altri investimenti. Addirittura apprendo dalla stampa che l'iniziativa è stata presa dalla ministra del turismo Daniela Santanché. Mi aspetto tanto quindi.

Stato per la cultura*. Signor Presidente, gentile senatrice Zambito, relativamente allo stato di ricostruzione del campanile della basilica di San Pietro Apostolo di Pisa, più nota con la denominazione di San Piero a Grado, risulta agli atti, quale ultimo progetto di ricostruzione finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali, quello redatto tra il 2005 e il 2007. I lavori, intrapresi alla fine del 2009, si sono arrestati al compimento del primo registro del campanile ad un'altezza di circa 15 metri. Il progetto, infatti, non risulterebbe oggi conforme all'intervento del decreto ministeriale del 17 gennaio 2018, che reca l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni. Pertanto, qualora fosse stabilito di riprendere la costruzione del campanile, andrebbe aggiornato il progetto o redatto un nuovo progetto. Negli ultimi cinque anni agli atti del Ministero non risulta alcuna richiesta di informazioni relative al campanile di San Piero a Grado e alla sua ricostruzione. Su invito dell'associazione «Amici dei musei» di Pisa, il 9 settembre 2022 si è compiuto un sopralluogo alla basilica di San Piero a Grado, insieme all'assessore all'urbanistica del comune di Pisa di Pisa e alla presidente della citata associazione, in occasione del quale proprio la presidente dell'associazione ha esposto la rinnovata attenzione al tema della ricostruzione del campanile; tema subito accolto con immediata disponibilità da parte degli uffici competenti nel valutare in quali termini tecnici e culturali potesse proporsi la ripresa della costruzione. A distanza di ormai ottanta anni dalla perdita dell'originario campanile si è subito espressa l'opportunità di interrogarsi prioritariamente sulle modalità di un'eventuale ricostruzione e di valutare, con la necessaria riflessione critica, l'eventuale declinazione esecutiva dell'ormai lontano principio del come e dove era. Con tale intendimento, nei primi mesi del 2023, la Soprintendenza ha promosso un incontro pubblico tra tutti gli enti direttamente coinvolti - Arci diocesi di Pisa, comune di Pisa e Soprintendenza e associazioni e comitati - ampliando il confronto anche alle istituzioni accademiche, realizzando una giornata di studio dal titolo "Danni di guerra e restauro dei monumenti": il caso del campanile di San Piero a Grado a Pisa. In tale occasione sono state registrate immediate adesioni della Scuola Normale Superiore di Pisa e di docenti, professori ordinari di restauro architettonico di varie università italiane, nonché della *ex* direttrice dell'Istituto centrale per il restauro. Tuttavia, la proposta avanzata da questa Soprintendenza non ha avuto esito. Inoltre, è opportuno precisare che gli uffici competenti del Ministero non hanno ricevuto alcuna richiesta, né relativi finanziamenti, con riferimento più in generale al tema della ricostruzione del campanile. In merito al danneggiamento della copertura della Basilica a seguito della caduta di un fulmine, avvenuta lo scorso 18 agosto, il giorno successivo la Soprintendenza di zona ha effettuato un sopralluogo, congiuntamente al personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Accertate le condizioni di degrado degli elementi lignei e di copertura e le conseguenti condizioni di pericolo, gli uffici nell'immediato e con urgenza hanno disposto l'affidamento dei lavori. A oggi risultano completati i ponteggi di lavoro e le puntellature necessarie a garantire la conservazione del bene e sono in corso di esecuzione indagini preliminari all'esecuzione degli interventi restaurativi. I lavori sono regolarmente tuttora in corso e si ritiene opportuno segnalare che sua eccellenza, monsignor Benotto, Arcivescovo di Pisa, ha espresso direttamente il proprio personale ringraziamento per l'immediato avvio dei lavori di urgenza con sua nota dello scorso 1° settembre.

ai senatori e al Sottosegretario, che lo sa senz'altro, quanto sia importante questo bene architettonico, e non tanto perché si trova a Pisa, nella mia città, ma perché è una Basilica romanica costruita nell'undicesimo secolo sui resti di un tempio paleocristiano. È attrazione per molti turisti durante l'anno ed è veramente un carattere distintivo della città di Pisa, della Toscana tutta e direi dell'intera Nazione. Per quanto riguarda il campanile, che è rimasto distrutto nel 1944, durante la guerra, molti progetti si sono susseguiti e alcuni sono stati finanziati. Tuttavia, dal 2008 in poi, non abbiamo più riscontrato alcuna attività

indignati e anche preoccupati perché, in realtà, molti progetti si erano susseguiti e molte idee erano state presentate all'amministrazione. Quindi, non riuscivamo a capire e capacitarci del motivo per cui l'amministrazione comunale, nonostante tutti gli impegni, convegni

Apprendere oggi che effettivamente corrisponde al vero che non vi è stata alcuna attività da parte di questa amministrazione per tentare di riportare agli antichi fasti la Basilica di San Pietro dispiace enormemente. Risulta anche a me - l'ho appreso soltanto dopo aver scritto questa interrogazione - il tempestivo intervento della Soprintendenza di Pisa e Livorno per ripristinare e mettere in sicurezza la Basilica dopo l'incendio dell'agosto scorso. È chiaro che mettere in sicurezza non vuol dire ripristinarla e, quindi, serviranno ulteriori interventi. Quindi, certamente non posso dirmi soddisfatta non per quello che ha risposto oggi il Sottosegretario. Non sono soddisfatta principalmente perché tutti i progetti che sono stati presentati al Comune di Pisa non sono mai stati finanziati, perché al Comune di Pisa nessuno si è degnato di chiedere il finanziamento al Ministero, e questo mi pare grave. Sono soddisfatta del fatto che si sia intervenuti tempestivamente, ma certo non sono soddisfatta del fatto che oggi non ho appreso da lei, Sottosegretario, se sono stati stanziati ulteriori fondi, non tanto per i progetti che non ci stanno e che il Comune non ha presentato, ma per ripristinare l'interno della basilica, non il campanile, in seguito all'incendio

Presidente, voglio portare in quest'Aula l'urgenza di ore che sono molto pesanti, anche drammatiche, per migliaia di lavoratrici e di lavoratori di uno dei settori industriali più nevralgici del nostro Paese, la cosiddetta filiera del "bianco", il settore dell'elettrodomestico italiano. È un settore portante dell'eccellenza del *made in Italy*, una filiera industriale storica e importantissima per il nostro Paese. Ebbene, ieri in un tavolo al Ministero

(c'erano i Sottosegretari, ma non c'era il Ministro e ci chiediamo dove fosse in un momento tanto decisivo), ha presentato un piano industriale che è devastante: un piano di chiusure e di licenziamenti che significherebbe la desertificazione industriale di interi territori. Secondo questo piano, dovranno chiudere entro il 2025 le fabbriche di Comunanza e di Siena nella loro totalità, così come il centro di sviluppo e di ricerca di Fabriano, dovrà essere ridimensionato pesantemente il nucleo di Cassinetta a Varese tagli al centro ricambi di Carinaro a Caserta. Un piano che prevede un totale di licenziamenti di oltre 2.000 lavoratori su un totale di 4.000 occupati, Presidente. Conosco molti di loro, le loro storie e delle loro famiglie. Conosco alcuni di questi stabilimenti: parliamo di professionalità, vite e lavoro che vengono cancellate di colpo, con una parola - "ristrutturazione" che è un inganno e un insulto, che in realtà è la volontà di andarsene dall'Italia. Noi diciamo no; non si può cancellare la storia di intere generazioni di operai e di tecnici, non si può cancellare la storia di interi territori che hanno contribuito a fare dell'Italia una potenza industriale. dove sia il Governo Meloni in queste ore, cosa faccia e perché finora sia stato inerme mentre si compiva questo disastro. Il ministro Urso, in maniera anche baldanzosa, aveva detto che avrebbe utilizzato la *golden power*. Dove sta? Stava scherzando? Noi chiediamo che il Governo intervenga con urgenza e con forza, facendo leva su tutte le sue prerogative, per impedire quella che sarebbe una catastrofe industriale e sociale colossale. Una crisi industriale, Presidente, mi lasci dire anche questo, che colpisce le aree del sisma del 2016. Non potrà esserci vera ricostruzione, se non si garantisce il mantenimento del tessuto produttivo locale. Per questo chiediamo un'informativa urgente in Parlamento non solo del ministro Urso, ma anche della presidente Meloni, perché c'è in gioco il futuro industriale dell'Italia. Servono investimenti, serve un progetto industriale vero, di rilancio rilancio dell'occupazione. Chiediamo al Governo risposte. Proprio in queste ore, adesso, in tutte le sedi ci sono presidi dei lavoratori. Noi siamo dalla loro parte. Penso che tutta questa Assemblea debba essere dalla loro parte. Continueremo a far sentire in quest'Aula la loro voce.

Signor Presidente, devo qui denunciare e segnalare quanto sta accadendo in queste ore e quanto è accaduto in particolar modo nella giornata di ieri presso l'università La Sapienza di Roma. Studenti di Azione universitaria, il gruppo universitario presente con i propri eletti in quella e in tutte le altre università italiane,

È una vicenda gravissima, che pone problemi molto seri, innanzitutto dal punto di vista della tenuta democratica e della garanzia democratica di poter esprimere le proprie idee. I collettivi e gli ambienti riconducibili ai collettivi e ai centri sociali di estrema sinistra ci fanno ripensare - ne parlavamo ieri con il presidente della 1a Commissione Balboni - a quella frase di Mino Maccari che diceva che il fascismo si divide in due parti: il fascismo propriamente detto e l'antifascismo. Certo antifascismo, l'antifascismo dei centri sociali e dei collettivi, ci ricorda proprio quella frase, perché l'antifascismo di chi affibbia l'etichetta di fascista a chiunque la pensa diversamente e si arroga il diritto di decidere se può entrare o meno nella città universitaria, se può o meno dare un volantino, se può o meno addirittura svolgere le proprie

delle elezioni, contrariamente a quanto di fatto sta avvenendo. Poi c'è anche un tema di allarme serio per il ritorno e per il crescere di un certo atteggiamento di violenza politica da parte dell'estrema sinistra, che va condannato e sul quale tutte le forze politiche dovrebbero essere unite, perché ricordiamo molto bene la lezione del passato e ricordiamo che i cattivi maestri, come oggi può essere un certo signor Raimo o altri, che fanno appello e che in qualche modo portano avanti un linguaggio di violenza,

politica. Una storia che non deve mai più tornare. Quindi fermiamoci, si fermi chi usa questo linguaggio e condanniamo tutti quanto accaduto alla Sapienza, perché non è tollerabile che dei ragazzi non possano svolgere le proprie iniziative e non possano addirittura fisicamente entrare dentro un'università, il cui accesso agli studenti deve essere garantito sempre e in ogni giornata.

alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro per lo sport

finestra") *(IV-C-RE)*. Signor Ministro, in un celebre film, uno dei miei preferiti di Massimo Troisi, «Le vie del Signore sono finite», ad un'esaltata amica della protagonista che sottolineava che da quando c'era lui - lui inteso come il duce - i treni arrivavano sempre in orario, il protagonista Massimo Troisi le risponde dicendo che potevano farlo capostazione invece di capo del Governo. Forse è per evitare che a lei si faccia un'analoga battuta, ma da quando c'è lei i treni non arrivano veramente neanche per caso o c'è un chiodo che blocca il Paese e lo divide in due, o addirittura per l'ansia del ritardo fanno partire cinquanta minuti prima i treni. E questo è successo a Genova: un treno doveva partire alle ore 16,20, ma la anticipata di cinquanta minuti, per la gioia dei passeggeri che si sono trovati senza treno. Non va meglio se uno decide di andare in aereo, perché c'è sempre una tratta intasata o un vettore vettore in ritardo e che deve essere allestito. Morale della favola, il 24 dicembre inizia il Giubileo e, quindi, forse bisognerà rivolgersi all'Altissimo perché finalmente le infrastrutture in questo Paese funzionino. Treni ed aerei

di prendere l'aereo invece del treno riuscirebbe ad arrivare puntuale. Insomma la fotografia del nostro Paese non è molto esaltante. *(Applausi)*.

Governo. In relazione al trasporto ferroviario, le cause dei disservizi da lei segnalate sono di diversa natura. I dati forniti dal gestore, che tengono conto di tutte le cause di ritardo, registrano una puntualità pari al 74

come estranei in linea, suicidi, eventi meteo rilevanti e altri fattori esogeni, incidono - ahimè - per una quota assolutamente preponderante, pari al 22 per cento sulle frecce, al 15,4 sugli intercity e al 6,6 sui regionali. Non possiamo sottostimare ovviamente il tema dei cantieri mai aperti numerosi come oggi: 1.200 cantieri e 9 miliardi di euro investiti solo nel 2024, cifra che non ha precedenti nella storia. Potrei chiudere un po' di cantieri, ma poi ne pagherebbero le conseguenze i nostri figli, fra qualche anno. Per contenere l'impatto di questi fattori di ritardo con azioni correttive, il gestore di infrastruttura ci segnala l'adozione di più misure di prevenzione e gestione delle emergenze, come il presidio *in loco* del personale, specifici piani di contingenza per fronteggiare ripercussioni, e di recente Trenitalia si è dotata di venti locomotive di soccorso diesel elettriche di ultima generazione, ad esempio. In relazione al trasporto aereo, ricordo che i disservizi causati dai problemi tecnici riscontrati quest'estate sono legati a problemi comuni ad altri Paesi europei. In termini numerici, infatti, nel periodo gennaio-settembre 2024 il traffico aereo in Italia ha registrato una crescita dell'11 per cento. Nonostante tale incremento, i tassi relativi ai disservizi restano circoscritti. Le cancellazioni, infatti, nei primi nove mesi del 2024 sono dell'1,1 per cento e i ritardi superiori alle due ore del 2,7 per cento. Per entrambe le tipologie di servizi, larga parte degli eventi è riconducibile al traffico internazionale. Sulla base di questi dati, ENAC ha avviato una ricognizione della capacità oraria dei singoli aeroporti. Ricordo infine che, anche in previsione dei grandi eventi da lei citati come il Giubileo e le Olimpiadi Milano-Cortina, ho personalmente attivato presso il Ministero un tavolo permanente con tutti gli operatori del settore per prevenire ulteriori disservizi e individuare le misure idonee a garantire la qualità dei servizi. È chiaro che con il *record* storico di investimenti e di cantieri aperti dei disagi ci possono essere. Mi spiace che questi cantieri e questi investimenti non li abbiano fatti coloro che c'erano prima di me.

dire - apprezziamo l'autocritica. Però, siccome prima di questo Governo c'era sempre lei al Governo, è complicato trarre un giudizio da ciò. L'unico *record* che lei ha conseguito è quello di un Paese di cui parlano tutti per i ritardi continui di tutti i mezzi di trasporto. Ecco il *record* che lei ha ottenuto in questi anni di Governo. Peraltro, i dati che ha dato in modo svogliato e semplicistico, come fosse una persona ormai chiusa dentro la torre d'avorio, che non si misura più troppo con il popolo, lo hanno in qualche modo dimostrato. Solo lei può spiegare agli italiani in diretta televisiva che i treni sono tutti in orario, che il gestore le ha comunicato che i treni sono in orario.

l'altra volta, per evitare che qualcuno vi contestasse il fatto che un treno arrivava in ritardo, avete fatto partire cinquanta minuti prima il convoglio nella direzione di Genova che - come sa - ha qualche problema di carattere infrastrutturale ancora non risolto. Se è vero che lei non è responsabile di quanto è accaduto, ci vuole dire se vuole far dimettere i vertici che sono attualmente a capo di RFI e di Trenitalia?

sulle ripercussioni degli scioperi nel settore dei trasporti di Salvini c'era anche lei al Governo, quantomeno con il Governo Draghi e anche con il Governo giallorosso, e forse i Ministri alle infrastrutture erano la De Micheli e prima ancora il ministro Toninelli. Quindi, se c'è una correità, questa c'è da parte di tutti, e non solamente del ministro Salvini. Salvini. Venendo all'interrogazione in oggetto, il diritto allo sciopero, sancito dall'articolo 40 della Costituzione, ha un rilievo fondamentale nella nostra società. Esso consente a tutti i lavoratori di affermare e rivendicare diritti e condizioni migliori sul lavoro. Tuttavia, anche il diritto dei cittadini di usufruire di un sistema di mobilità pubblica trova tutela costituzionale, in particolare alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 16, 33 e 34. Il trasporto pubblico, infatti, offerto a condizioni accessibili a tutti, consente di neutralizzare le disparità sociali e di conferire uguali opportunità di lavoro e d'istruzione ai cittadini meno abbienti, che non sempre possono sostenere il costo della mobilità privata per recarsi sul luogo di lavoro o per raggiungere l'istituzione scolastica o universitaria. Le rivendicazioni in termini di migliori condizioni e sicurezza dei lavoratori del settore dei trasporti sono giuste e condivisibili. E il Governo e questa maggioranza hanno già cominciato a intervenire con misure *ad hoc*, ad esempio in tema di sicurezza a bordo di treni Tuttavia, la quantità di scioperi nel settore dei trasporti proclamati negli ultimi due anni ha assunto dimensioni inedite, manifestandosi, soprattutto in alcune città, con cadenza periodica mensile e, talvolta, settimanale. In tali circostanze, per svolgere qualsiasi attività abituale, quale ad esempio recarsi sul posto di lavoro o semplicemente portare i propri figli a scuola, i cittadini sono costretti a riorganizzare le proprie abitudini e, in particolare, chi usufruisce quotidianamente del trasporto pubblico deve necessariamente servirsi di mezzi privati. Ciò provoca sicuramente sicuramente forti disagi alla mobilità, ma anche gravi danni ambientali, a causa degli elevati valori di agenti inquinanti che vengono immessi nell'aria nelle ore di punta per l'utilizzo obbligato di auto private. Si chiede di sapere quale quale sia la consistenza degli scioperi di settore proclamati negli ultimi due anni e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per garantire sicurezza e condizioni migliori per i lavoratori del settore e, allo stesso tempo, per salvaguardare il diritto di tutti i cittadini di usufruire del sistema di mobilità pubblica per le fondamentali esigenze di

sono stati proclamati 518 scioperi nazionali e interregionali, di cui 374 realmente effettuati, per una media di 15 scioperi al mese. Facendo un confronto con i Governi precedenti, si tratta della media mensile più alta degli ultimi sette Governi. Evidenzio, ad esempio, che, durante i trentaquattro mesi del Governo Renzi, i sindacati erano più distratti, perché gli scioperi furono 280, per una media di quasi la metà di quelli di oggi. Tra gli scioperi più impattanti, segnalo 57 scioperi nazionali e interregionali effettuati nel settore ferroviario, a fronte dei 71 proclamati, e 34 scioperi nel trasporto pubblico locale sui 39 proclamati, di cui la maggior parte svolti nei giorni di lunedì e venerdì. Sono dati che inducono a una riflessione sulle ragioni del ricorso a un istituto fondamentale per la tutela dei lavoratori, così come sul relativo impatto sugli utenti. Ritengo sia assolutamente legittimo rivendicare salari migliori e più sicurezza, e su questo stiamo lavorando anche in questa legge di bilancio. Sono temi su cui il Governo ed io personalmente ci stiamo impegnando. Pertanto, auspico che i sindacati possano con senso di responsabilità rivalutare le modalità degli scioperi programmati nelle prossime settimane per garantire il diritto al lavoro, alla salute e allo studio di milioni di cittadini italiani incolpevoli. Tra le iniziative promosse dal MIT, segnalo che è stato riattivato il tavolo previsto dal protocollo per la promozione della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale e regionale. Rispetto alle misure di potenziamento della sicurezza dei lavoratori e degli utenti del settore trasporti, ho provveduto a emanare il decreto ministeriale per l'installazione sugli autobus di paratie di protezione per i conducenti e di dispositivi che consentano la geolocalizzazione e la chiamata di emergenza alle Forze dell'ordine. Con specifico riferimento al tema della sicurezza nel settore ferroviario, evidenzio che dall'avvio dell'attività della società FS security, nata nel 2023, in coincidenza con l'avvio di questo Governo, sono stati incrementati i controlli sui viaggiatori e, a bordo dei treni, è stata anche avviata la sperimentazione con la fornitura di *bodycam* agli addetti del controllo a bordo (1.100 donne e uomini in pettorina che chi prende il treno vede in stazione e sul treno). Ricordo inoltre che, per assicurare la sicurezza nelle stazioni, con la legge di bilancio 2025 abbiamo previsto anche la proroga del contingente previsto per l'operazione «Stazioni sicure» fino al 2027. In conclusione, i numeri mi sembrano chiari; mai stati così tanti scioperi come contro questo Governo, qualcuno invita alla rivolta sociale. Se gli scioperi vengono svolti rispettando le norme, *nulla quaestio*; altrimenti, già dalle prossime ore, interverrò personalmente per limitarne la fascia oraria, eventualmente anche con la precettazione.

trovato nei periodi precedenti il suo mandato treni puntuali; sicuramente avevo trovato stazioni con meno presenza di polizia e servizi a garanzia della sicurezza Lei, Ministro, ha fatto molto bene a rivendicare il tema della legittimità e la necessità di avere salari più alti e una maggiore sicurezza. Ha anche elencato quelle che sono le misure già intraprese da questo Governo attraverso il suo Ministero. il suo Ministero. Sul tema della sicurezza lei ha ben specificato la questione legata alla FS security, con la possibilità della *bodycam* e il fatto di avere più personale nelle stazioni. Faccio riferimento a un evento accaduto ieri nella mia provincia: una persona a bordo di un treno trovata senza biglietto è andata in escandescenza; il controllore ha dovuto chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine. La persona è stata arrestata perché ha tirato un pugno a un poliziotto. Questa persona della Sierra Leone, con diversi precedenti in tal senso, è stata arrestata. arrestata. Questa è la situazione che abbiamo ereditato grazie a una politica delle porte spalancate a tutti, di cui oggi noi andiamo a pagare le conseguenze. Certamente non favoriscono il lavoro della polizia quei giudici che il giorno dopo rimettono in libertà soggetti socialmente pericolosi.

Siamo riusciti, anche con il suo aiuto, a definire quello che era il commissario nazionale per la brucellosi e la tbc, uno dei problemi che ha

la mozzarella - come ormai tutti sanno - è il primo formaggio per volumi in Italia, per un fatturato di 2008 miliardi di euro l'anno, con una crescita del 9,33 per cento. In questi momenti, Presidente, può comprendere che sarebbe uno dei comparti da favorire quanto possibile. La legge possibile. La legge del 2014 tutelava i trasformatori e i produttori della filiera bufalina, ma anche la trasformazione della mozzarella.

invaso da latte e da cagliata di latte di bufala estera non tracciata, consentendo così ai caseifici e alle cooperative di riempire le celle frigo con la conseguente disdetta dei contratti firmati con i produttori, il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato e come intenda intervenire per potenziare l'efficacia attuativa delle norme citate a tutela della tracciabilità del latte di bufala, anche valutando la possibilità di costituire un organismo centrale con ruolo di controllo e di indirizzo; se intenda promuovere l'adozione di un piano triennale di monitoraggio verifica e il controllo incrociato tra il latte e le cagliate di latte di bufala prodotto ovvero introdotto in Italia, e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP e quella della mozzarella di latte di bufala generica, prevedendo verifiche periodiche nelle piattaforme, relativamente alla veridicità dei dati inseriti, e nelle strutture frigo di stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione,

di bufala campana DOP e un comparto che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare importanti criticità legate all'incremento dei costi produttivi e alla diffusione di patologie animali, come la brucellosi. In questo difficile scenario il Governo Meloni è al fianco delle aziende in un percorso di rafforzamento della filiera e di valorizzazione del prodotto a livello nazionale e internazionale. Con la nomina di un commissario straordinario, che lei ha ricordato essere stato frutto del lavoro congiunto tra Parlamento e Ministeri - è infatti il Ministero della salute il Ministero della salute ad avere responsabilità su questo tipo di situazioni - si è attivato un processo che riteniamo migliorativo dell'azione per contrastare la piaga della brucellosi e della TBC anche negli allevamenti bufalini. Fenomeni fraudolenti come quelli denunciati dall'interrogante rappresentano fatti di estrema gravità che rischiano di ostacolare questo percorso di crescita, andando a ledere l'immagine di eccellenza della mozzarella di bufala e danneggiare la stragrande maggioranza degli operatori che agiscono - questo va sempre chiarito - nel rispetto delle regole e della tradizione. Per l'azione di contrasto abbiamo potenziato il Comando dei carabinieri per la tutela agroalimentare, il CUFA, e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, proprio al fine di garantire la massima efficacia e capillarità delle operazioni di controllo nel settore agroalimentare. Inoltre, andando incontro a un'esigenza che lei ha richiamato, abbiamo creato una cabina di regia interforze, istituita lo scorso anno, che coinvolge anche l'Agenzia delle dogane, l'AGEA, la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza per evitare le importazioni fraudolente che tanto danneggiano. È proprio in sede di cabina di regia per i controlli agroalimentari che, nella seduta dell'8 agosto 2024, è stata esaminata la problematica dei controlli sulla tracciabilità del latte bufalino ed è stata assunta la decisione di intensificare l'attività di contrasto alle pratiche illecite. È un dato significativo che, nei primi dieci mesi del 2024, l'Ispettorato della tutela della qualità abbia già realizzato 441 controlli ispettivi sulla filiera di latte di bufala, andando oltre i 382 controlli realizzati nel 2023. Ulteriori 46 ispezioni sono state eseguite quest'anno dal Comando dei carabinieri per la tutela agroalimentare ed altre sono programmate nei prossimi giorni, unitamente al personale ispettivo dell'ICQRF. Tali controlli riguardano la tracciabilità e le giacenze fisiche e contabili del latte bufalino, dei semilavorati e delle produzioni DOP e non DOP, anche al fine di riscontrare la provenienza delle materie prime utilizzate. Nel contempo, stiamo avviando un percorso di miglioramento della piattaforma informatica del latte di bufala, istituita a partire dal 2014 all'interno del SIAN, in collegamento con la banca dati dell'istituto zooprofilattico di Portici, al fine di ottimizzare i meccanismi di verifica dei quantitativi di latte presente nei caseifici e la sua destinazione produttiva, anche in collaborazione - ovviamente - con il Ministero della salute. Infine, annuncio che è in corso di elaborazione un disegno di legge collegato alla legge di bilancio, che il Governo presenterà nei primi mesi del 2025, volto a rivedere il sistema sanzionatorio in materia agroalimentare e nel quale abbiamo intenzione

che in questa risposta è stato abbastanza chiaro nel dire che esiste una sinergia tra le varie forze in campo, che non c'è quindi questo comparto stagno dietro al quale nascondersi nel dire che non è sua competenza. Per quanto riguarda la mozzarella di bufala DOP campana, significa parlare di un indotto, significa parlare di tutela dell'origine, visto che il disciplinare dice in maniera prioritaria che il latte debba essere di provenienza casertana. casertana. Quindi significa tutelare i produttori di latte, gli allevatori: un indotto. Significa dare opportunità di lavoro, significa anche tutelare l'occupazione, il cambio generazionale, dare quindi fiducia anche ai giovani in quella che può essere un'opportunità lavorativa importante. A me dispiace che non sempre c'è questa voglia di entrare in quello che non è vero che non è sua competenza personale. Io volevo presentare un'interrogazione per quanto è stato rappresentato nel programma «Report», ma non mi è stato concesso di presentare a lei l'interrogazione, perché dice che tutto quanto è emerso in quel servizio non è di sua competenza. Nel decreto agricoltura abbiamo rifinanziato il fondo per quanto riguarda gli interventi strutturali e funzionali per la biosicurezza, ben 5 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025: biosicurezza che deve essere controllata proprio da lei, perché non penso che i fondi stanziati, penso che i fondi stanziati, che provengono dalle tasse dei cittadini, debbano essere buttati dalla finestra senza un controllo. Il commissario stesso non può agire, ma segue le può agire, ma segue le indicazioni del Ministero. Quindi, auspico questo lavoro di squadra e questa sinergia, perché altrimenti siamo rovinati. Anzi, da oggi in poi vorrei che lei, Ministro, in prima persona segua tutto il discorso e dia fiducia ai produttori. E soprattutto non sprechiamo soldi quando poi i danni da rincorrere e finanziare consisterebbero in centinaia di milioni di euro.

Signor Presidente, un breve inciso sulla replica della senatrice Naturale. Anche noi volevamo parlare di questo grave dramma della peste suina africana. Nella correttezza dei rapporti ci è stato detto che non era di esclusiva competenza del Ministero dell'agricoltura, però oggi vogliamo dire che questo è un tema che qualcuno deve affrontare al Governo, perché ne va del lavoro di molti allevatori. L'allevamento è una competenza specifica dell'agricoltura. Comprendiamo anche che le epidemie possono essere di competenza di altri Ministeri, Ministeri, ma non si può fare una melina tra un Ministero e un altro. È necessario che al Paese, agli italiani, ai produttori, agli agricoltori e ai parlamentari siano dati i giusti strumenti per aprire una discussione su un tema estremamente essenziale. Attualmente giacciono tre interrogazioni in 9a Commissione

Per contro c'è un aumento della domanda, legata soprattutto al grano duro per quello che attiene ai pastifici, a questa industria particolarmente identitaria del nostro Paese; ma ciononostante i prezzi

perché la semina avviene in questo periodo. Molti agricoltori non si sentono più in grado di sostenere i costi di produzione, che ormai sono arrivati a circa 1.100 euro a ettaro, quando se ne ricavano circa i due terzi dalla vendita del grano stesso. Con la nostra interrogazione chiediamo al Ministro quali sono le misure che il Governo intende assumere, anche alla luce dell'inefficacia di alcuni interventi fatti con il decreto agricoltura, e quali sono le prospettive che si individuano per questo settore. Signor Presidente, lo dico sia al collega Franceschelli, sia alla senatrice Naturale: io rispondo sempre alle domande che mi sono proprie. Conoscete il Regolamento del Senato: non spetta a me determinare quali sono le cose a cui posso rispondere. Se si pongono quesiti al Ministro dell'agricoltura che riguardano le sue competenze, può rispondere lui; altrimenti deve rispondere un altro collega. Sono ben pronto, però, a dare la mia massima disponibilità a rispondere a qualsiasi quesito in qualsiasi circostanza, nei modi e nei tempi dovuti e con il rispetto dei Regolamenti delle Aule che ci ospitano. Ringrazio il collega Franceschelli, perché ha posto l'attenzione su un settore vitale per l'agroalimentare italiano, quella cerealicolo. C'è davvero un'emergenza complessiva rispetto ai prezzi e rispetto all'elemento deficitario e alla carenza strutturale di produzione nella incrementata per avere quella sovranità alimentare che prima sembrava cercasse solo l'Italia e che oggi tutta l'Europa e probabilmente gran parte del mondo ritengono una priorità. Mi preme innanzitutto rilevare che il Ministero dell'agricoltura segue con estrema attenzione le questioni che afferiscono al settore cerealicolo, una delle filiere più fragili e al contempo strategiche per il *made in Italy* agroalimentare. Per tale motivo sono molteplici gli strumenti messi in campo dal Ministero a sostegno della coltura cerealicola e a supporto della produzione nazionale. Innanzitutto, la politica comune della PAC garantisce un sostegno al reddito attraverso i pagamenti diretti per assicurare un'adeguata remunerazione al settore cerealicolo; anche l'efficientamento dei tempi va incontro alle esigenze degli imprenditori agricoli. In particolare, la filiera del grano duro è sostenuta con il pagamento accoppiato per le aree del Sud Italia, con risorse pari a 93 milioni di euro l'anno. Sul fronte nazionale, siamo intervenuti più volte a sostegno della filiera del grano duro e del comparto cerealicolo più in generale. Innanzitutto desidero rammentare l'istituzione del Fondo per la sovranità alimentare, destinato a dare sostegno alle filiere cerealicole del mais, dell'orzo e del frumento tenero, che non rientravano tra quelle sostenute sostenute dalla PAC, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro fino al 2026, incrementata con ulteriori 11 milioni di euro dal decreto-legge agricoltura, che lei richiamava. Successivamente, a seguito della crisi che ha investito il settore del grano duro, abbiamo stanziato per il 2024 risorse pari a 32 milioni di euro, di euro, raddoppiando il premio ad ettaro da 100 a 200 euro. Ulteriori risorse sono state stanziate per l'operatività della commissione unica nazionale (CUN) del grano duro, istituita da diversi anni, ma mai realizzata. Si tratta di uno strumento utile per una maggiore trasparenza e una più oggettiva determinazione dei prezzi. Lo stesso provvedimento ha garantito l'attivazione, a partire da gennaio 2025, di Granaio Italia, un innovativo ed efficace strumento di monitoraggio e trasparenza delle quantità e tipologie di cereali italiane ed estere presenti sul mercato nazionale. L'azione di Governo si è concentrata anche sulla tutela e sulla salvaguardia delle produzioni nazionali. A questo fine è stata istituita una cabina di regia,

procedura di selezione finalizzata all'individuazione di specifici progetti di ricerca; è l'altra sfida che dobbiamo raccogliere in maniera trasversale, per il miglioramento genetico dei cereali e per le innovazioni sulle quali poi investire per efficientare il sistema. In particolare, c'è stato un grande impegno trasversale di gran parte del Parlamento sulle tecnologie evolutive avanzate, superando i pregiudizi nei confronti di tecniche che ci possono mettere in condizione, come già avvenuto agli inizi del secolo scorso, di avere colture più produttive e più resistenti agli effetti del cambio climatico.

è chiaro che le misure messe in campo sono molteplici, ma non possiamo ritenerci soddisfatti; lo saremo solo quando il costo di produzione sarà inferiore al prezzo al prezzo di vendita, cioè quando gli agricoltori avranno la giusta remunerazione: questo è l'unico elemento che può contare. Chi amministra lo sa: io faccio anche il mestiere di sindaco e lei fa il mestiere di Ministro, e sappiamo che quando dobbiamo dare risposte ai cittadini, agli agricoltori, alle forze sociali, quelli che contano sono i fatti. Allo stato attuale il settore cerealicolo vive una crisi che potrei definire epocale, anche perché ci sono nuovi mercati che si affacciano, come quello della Turchia, mentre il mercato del Nord America è sempre stato molto forte. Vedremo anche quello che riuscirà a fare il Governo Meloni in Europa, perché oramai non si può nemmeno più dire che le politiche le facevano altri, vista anche la recente nomina del ministro Fitto. Diciamo pertanto che il panorama dell'analisi del passato è finito; ora c'è solo quello delle responsabilità e dei risultati, e la differenza lo farà solo questo. Concludo, signor Ministro, rivolgendole un appello per la sensibilità che ha per il mondo agricolo. In questi giorni è in discussione il decreto-legge sicurezza.

e il mercato che andremmo a perdere per una questione che nulla ha a che vedere con una produzione agricola e industriale andrebbe a vantaggio di altri Paesi e creerebbe ulteriori scompensi e perdite produttive nelle aree interne, quelle più deboli dove anche una piccola produzione può fare la differenza per la sopravvivenza di un'azienda.

Giornata mondiale della pesca e direi che è particolarmente pertinente questa interrogazione, a prima firma del senatore De Carlo. Quindi, sono ben felice di sottoporgliela conoscendo la sua sensibilità, attenzione, nonché efficacia nei confronti dei problemi dell'agricoltura, nel caso specifico della pesca, essendo comparto del settore primario. Premesso che la Commissione europea nel settembre 2024 ha adottato la Proposta sulle opportunità di pesca per il 2025 per il Mediterraneo e il Mar Nero, che approderà sul tavolo dei Ministri dell'Unione europea della pesca il 9 e il 10 dicembre per il via libera finale, tale provvedimento introdurrà delle misure che stabiliranno molto probabilmente limitazioni alle attività di pesca per il comparto ittico italiano, in termini di riduzione delle giornate di pesca. Ciò potrebbe comportare sensibili ripercussioni nel settore ittico, messo a dura prova anche dagli eventi climatici avversi che hanno colpito le coste italiane. Si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in sede europea affinché siano salvaguardati gli interessi delle imprese italiane e del settore della pesca. il senatore Amidei e il Gruppo Fratelli d'Italia, che ha presentato un'interrogazione che ci permette di trattare un tema strategico, come lei ha ricordato, in un giorno particolarmente importante. Oggi per la verità sono diverse le cose da ricordare:

purtroppo, il settore della pesca, per politiche nazionali, ma più che altro europee ha visto un tracollo insostenibile: meno 28 per cento delle marinerie europee, meno 40 per cento delle marinerie italiane. Un vero disastro che ci mette in condizione di invertire questa tendenza con fatti concreti.

ponga in maniera ineludibile la parola fine al declino della pesca, perché non siamo disposti a rinunciare in nessun modo a questo settore, ai benefici per il nostro nutrimento, ai benefici per l'ambiente (considerata la protezione del mare che i pescatori mettono in campo) e per i territori che ospitano le nostre marinerie, che vengono qualificati qualificati per mille ragioni dalla loro presenza. In Europa non sempre ci siamo trovati in buona compagnia. Abbiamo votato no anche da soli al Piano d'azione europeo sul divieto della pesca a strascico, perché è una pesca propria delle nostre marinerie e tale divieto metterebbe in ginocchio il nostro settore. La comunità scientifica, peraltro, è divisa sugli effetti di questa tipologia di pesca. Ciò vuol dire essere isolati in Europa? No, al contrario, in Europa abbiamo aperto la strada a una critica costruttiva nei riguardi di quello che era un modello ideologico che poneva in essere azioni che non venivano riscontrate nei risultati rispetto a quanto pianificato. Quello che chiediamo è dati scientifici e analisi di quello che avviene nel bacino del Mediterraneo (il nostro bacino principale); abbiamo denunciato che allo smantellamento delle nostre marinerie spesso, dall'altra parte del mare si contrappongano nuove barche che pescano senza regole, senza quel rispetto che invece i nostri pescatori hanno del patrimonio ittico. Il Governo italiano ha investito sulla pesca, ha modificato la legge n. 102 del 2004, una norma che era dedicata agli agricoltori quando venivano colpiti da eventi calamitosi, non era aperta ai pescatori. Oggi i pescatori sono messi sullo stesso piano e hanno ristori e rimborsi che permettono loro di superare criticità come quelle avvenute poc'anzi con l'aggressione del granchio blu all'acquacoltura, ma sono tante quelle che subiscono Abbiamo lavorato per maggiori controlli, perché bisogna raccontare e spiegare, sia in fase preventiva, sia in fase repressiva, che cosa avviene spesso in questo settore dove la qualità del nostro pesce viene messa in concorrenza con un pescato che ha meno controlli ed è meno salubre per la salute dei nostri cittadini. In Europa in ventiquattro mesi è cambiato l'approccio nei confronti di questi settori strategici; è tornata al centro la sovranità alimentare, cioè la ricerca dell'Europa di garantire, al di là delle contingenze, la possibilità di avere buon cibo e di trasformare, per continuare a essere Continente Continente esportatore. Ovviamente ci interessa il destino dell'Italia in primo luogo. Abbiamo lavorato in questi giorni, proprio nell'ultima Agrifish, la riunione dei Ministri dell'agricoltura e della pesca, per redigere un documento unitario con la Francia e con la Spagna, seguiti poi da tante altre Nazioni, per chiedere una moratoria della riduzione forzata delle giornate di pesca, della riduzione senza dati scientifici dei contingenti di pescato.

oggi, grazie all'impegno della presidente Meloni in Europa e all'autorevolezza di questa Nazione, che dobbiamo ricordare essere protagonista in Europa, da sempre, fin dalla sua composizione, potrà coordinare anche i settori dell'agricoltura e della pesca. È cambiata la direzione dell'Europa, grazie a questa Nazione - l'Italia - che torna a fare il mestiere che la Storia le ha attribuito.

con cognizione di causa. Infatti ho avuto modo non solo di conoscere il ministro Lollobrigida per storie che ci appartengono di carattere politico e ideologico, ma l'ho visto alle prese con un problema quale il granchio blu. Io provengo dall'area interessata, il delta del Po', l'area di Chioggia e la zona di Goro. Immediatamente lei, Ministro, è intervenuto concretamente, non solo con la presenza fisica, stanziando subito Siamo nel distretto ittico più importante d'Europa, quello della vongola verace, quello della cozza DOP, quello dell'ostrica rosa, sono più che mai opportune ed ispirano grande fiducia per credere che effettivamente lei, come Ministro, possa dare delle risposte concrete

comunque il mestiere più antico del mondo e, anche da un punto di vista religioso, ha sempre rappresentato la speranza, la fiducia, il cibo, la continuità, soprattutto per i giovani, in un ricambio generazionale che nella pesca è particolarmente necessario.

è fondamentale per la conservazione e per il miglioramento della salute di ciascuno di noi. Negli ultimi decenni, la corsa ha avuto sempre più successo come modo popolare di mantenersi in forma e quindi di praticare sport nel proprio tempo libero, al di là, ovviamente, delle manifestazioni agonistiche di alto livello. Per questo, c'è stato un fiorire di eventi organizzati

piccolo gruppo di campioni che sono l'esempio per loro, ma poi la grande massa è fatta di persone che pagano per partecipare, che viaggiano per andare nel posto dove si fa questa gara e che portano un indotto importante per per molti territori. Ho fatto e faccio parte di comitati organizzatori, quindi so di che parlo. A questo riguardo, si pone il tema della certificazione sanitaria. Ebbene, non si direbbe, ma trent'anni e 30 chili fa ho fatto la maratona di New York quella occasione compilai un modulo in cui attestai che ero a posto dal punto di vista sanitario, dovetti presentare anche il certificato di assicurazione e con quello venni iscritto. In Italia non è così: tuttora bisogna iscriversi presentando un certificato medico che ha caratteristiche specifiche per il nostro Paese, diverse da quelle che ci sono negli altri Paesi. Ciò comporta che in particolare quelli che vengono dall'estero hanno spesso delle difficoltà o che vi siano dei fraintendimenti e dei *qui pro quo* all'atto dell'iscrizione. La Federazione italiana atletica leggera ha provato a ovviare a questo tema facendo un regolamento in cui dà la possibilità di iscriversi come

del mio diplomino dove c'è scritto il numero del mio piazzamento e della foto ricordo del momento in cui taglio il traguardo. Il fatto che ci sia della gente che partecipa a gare di corsa senza entrare in classifica un *unicum* nel mondo. Credo che dobbiamo prendere atto che i cittadini hanno interesse essi stessi alla loro salute e che quindi non è che perché uno è chiamato a fare un'autocertificazione significhi che è pronto a certificare il falso. Chi fa sport normalmente si fa controllare e quindi auspico che anche in Italia si possa fare come all'estero, dove autocertificando di essere a posto con la salute si può partecipare a questo tipo di competizioni.

questa richiesta circa la mia posizione relativa ai requisiti di partecipazione in Italia alle manifestazioni sportive non agonistiche o di tipo ludico-motorio collegate alle attività su strada della Federazione italiana atletica leggera. Si tratta di un'interrogazione che mi consente anche di collegare in modo virtuoso nello spirito e nei contenuti l'articolo 32 e l'articolo 33 della Costituzione proprio relativamente al tema della tutela della salute e al diritto allo sport per tutti. Il Ministero della salute, a seguito del decreto 24 aprile 2013, ha emanato l'8 agosto 2014, integrandole nel 2015, le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, demandando al CONI il compito di distinguere i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate da coloro i quali svolgono attività sportive che non comportino impegno fisico, dai tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, obbligando solo i primi ad effettuare la visita medica. Il 10 giugno 2016 il CONI emanato una propria circolare, chiarendo con il parere favorevole del Ministero della salute, che l'obbligo di certificazione medica per la pratica di attività sportiva non agonistica è posto solo a carico dei soggetti tesserati che svolgono attività sportive regolamentate ovvero a carico dei tesserati che praticano un'attività sportiva non agonistica organizzata dal Coni, da società o associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva purché non si tratti di attività caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Da parte sua la Federazione italiana di atletica leggera al fine di agevolare la partecipazione a gare agonistiche organizzate sotto la propria egida di corsa su strada, *cross*, montagna e *trail* anche da parte di soggetti non tesserati ha istituito lo strumento denominato Tale strumento subordina la partecipazione dei sottoscrittori al possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per l'atletica leggera in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato anche digitalmente alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. A seguito delle linee guida del Ministero della salute e della circolare Coni, a partire dal 2021, la FIDAL ha introdotto anche un regolamento per le gare organizzate sotto l'egida della FIDAL stessa. Mi rendo conto che la sua richiesta va nella direzione di allargare una partecipazione che entri anche nell'ambito competitivo però, volendo sintetizzare per rimanere anche nei tempi, pur comprendendo lo spirito della sua proposta, ritengo che questa sua esigenza di semplificazione in qualche maniera, anche al fine di rendere il nostro Paese più competitivo nell'ambito dell'attrattività rispetto al turismo sportivo e alla partecipazione alle gare, debba necessariamente essere subordinato alla tutela della salute. Credo sia prioritario da questo punto di vista, ragionare su un allargamento ulteriore che consenta di poter competere e, quindi, di non partire nelle retrovie, cosa che la FIDAL sta già facendo di fatto. La priorità - ripeto ancora una volta - della tutela della salute si consolida anche attraverso lo sviluppo della cultura della prevenzione che ha nei controlli medici e nella relativa certificazione un elemento essenziale, anche quale patrimonio essenziale di informazioni che arricchirà l'identità digitale per la componente sportiva; un progetto che stiamo iniziando a elaborare con il dipartimento per la trasformazione digitale e l'innovazione tecnologica, guidato dal sottosegretario Butti, in collaborazione con la nostra società «Sport e salute». Stiamo cercando di contemperare le esigenze da lei segnalate con l'esigenza per noi prioritaria di salvaguardare la salute come bene primario. Come ho detto anch'io all'inizio, la salute è sicuramente fondamentale ed è la ragione per cui promuoviamo lo sport. Mi permetto di suggerire di guardare cosa fanno, ad esempio, in Francia, dove sicuramente non hanno meno a cuore la salute di quanto non l'abbiamo a cuore noi, ma consentono di partecipare senza bisogno di presentare fisicamente un certificato medico. Ho la sensazione, Ministro, che il problema è una mentalità istituzionale italiana; quando qualcuno controllare se l'organizzatore ha nella fila dei suoi certificati medici anche quello lì e sia in ordine, invece che andare poi a verificare da ogni singolo che dovesse avere dei problemi di salute se è a posto dal punto di vista dei controlli e della prevenzione. Capisco, però bisogna anche cominciare ad avere fiducia nei cittadini e a non ribaltare sempre sugli organizzatori, che fanno oggettivamente fatica a svolgere questo ruolo, la responsabilità della verifica dello stato di salute di coloro che partecipano alle loro gare. La ringrazio in ogni caso.

Signor Presidente, ministro Abodi, i senatori di Forza Italia hanno predisposto un disegno di legge per rinnovare e accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli stadi con l'obiettivo principale di modernizzare le infrastrutture, semplificando le procedure burocratiche e favorendo gli investimenti privati. La nostra proposta prevede che i permessi per i lavori vengano rilasciati in tempi brevi, in modo simile alle ZES, che stanno funzionando molto bene, per rispettare i tempi di realizzazione degli impianti. Per incentivare gli investimenti abbiamo previsto anche un credito d'imposta per i progetti sostenibili. La nostra proposta ha l'ambizione di trasformare gli stadi in centri multifunzionali di aggregazione sociale, culturale e sportiva. Ogni progetto dovrà includere un piano urbanistico in modo da contribuire a rigenerare anche le aree circostanti e sarà inoltre necessario ricorrere a concorsi per i progetti internazionali per garantire elevati livelli di *standard*.

Il piano punta su sostenibilità, innovazione e valorizzazione del patrimonio impiantistico calcistico. Si tratta di un tema che porterà vantaggi soprattutto al Sud Italia, dove la maggior parte degli impianti sono stati realizzati più di sessant'anni fa (quindi oggi si trova all'interno dei nuovi perimetri urbani). quindi rigenerare parti importanti di città. Lo scopo è dotare le nostre città di impianti sportivi all'avanguardia, ma non solo, anche di poli che possono diventare multifunzionali e di aggregazione dal punto di vista sociale e culturale. Le chiediamo, Ministro, la sua posizione sul tema della necessità di avere queste infrastrutture sportive come stadi più moderni e integrati nel tessuto cittadino e se ha in mente o ha avviato iniziative in questo senso.

del Ministro e del Governo su questa tematica, peraltro in continuità con le linee di indirizzo che ho espresso all'inizio del mio mandato. Ciò al fine di spiegare, all'interno delle politiche sportive, il ruolo centrale, o comunque significativo e strategico, dello sviluppo di tutte le infrastrutture, con particolare rilievo per quelle sociali (quindi quelle di base) e per quelle, per quanto altrettanto sociali, più sofisticate dal punto di vista industriale, ovvero gli stadi. Possiamo saltare i preamboli perché questo tema è stato trattato ormai da decenni e siamo rimasti molto indietro rispetto al resto dell'Europa soprattutto, e del mondo. Andiamo quindi al cuore della questione. Ringrazio non soltanto per questa interrogazione, ma anche per lo schema di disegno di legge che avete presentato, che si inserisce nell'ambito delle attività che abbiamo già posto in essere come Governo, soprattutto nell'ambito delle deleghe che mi sono state affidate. Al Ministero dell'economia e delle finanze è stato costituito un gruppo di lavoro permanente con il ministro Giorgetti e tutta la struttura tecnica dei rispettivi Ministeri, al quale partecipano i vertici tecnici di CDP, Invimit, SACE, l'Istituto per il credito sportivo e culturale e Sport e Salute. Questo gruppo di lavoro ha un obiettivo preciso: in tempi molto brevi elaborare un portafoglio di opportunità finanziarie che non prevedano fondo perduto, ma comunque agevolazioni in termini di *equity,* garanzie e contributi in conto interessi e che propongano semplificazioni ulteriori che ci riproponiamo di inserire in una legge delega che è in via di predisposizione e che segue al correttivo del decreto legislativo n. 38 del 2021 che abbiamo approvato lo scorso anno, il quale semplifica l'*iter* amministrativo, adeguandolo anche alle nuove norme del codice dei contratti, e facilita anche le compensazioni industriali e commerciali, delocalizzandole rispetto agli stadi. Abbiamo già iniziato da sei mesi un confronto serrato con le amministrazioni comunali e con i *club*, proprio perché vogliamo dare un calendario che dia il senso del tempo che è passato e del poco tempo che abbiamo avanti per ammodernare il patrimonio immobiliare, in gran parte pubblico, che è rappresentato dagli stadi, la cui evoluzione rappresenta uno strumento formidabile di riqualificazione e rigenerazione urbana, caratterizzato dall'accessibilità, dall'intelligenza tecnologica, dall'educazione ambientale e dalla funzionalità. Lo abbiamo iniziato a fare con le amministrazioni e i *club* per gli stadi di Bologna, Firenze, Cagliari, Empoli e Parma e proseguiremo con Verona, Genova, Napoli, Palermo e Milano, non soltanto con l'obiettivo di arrivare competitivi alla selezione degli stadi per Euro 2032, quanto per la necessità, comunque, di essere competitivi nella logica del miglioramento dell'offerta sportiva dedicata al pubblico. Lo stadio infatti è fatto per essere frequentato in modo civile, adeguato e partecipato, soprattutto

che sono state svolte, nell'ottica di una proposta che riguardi il sistema calcistico nella sua complessità, convinti che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Signora Ministro, non avevamo dubbi sul fatto che lei e il Dicastero da lei guidato foste favorevoli ad investire negli impianti sportivi e negli stadi in particolare, perché lo stadio - come più volte lei ha ripetuto - è un sistema produttivo, ma anche un un centro di aggregazione sociale con risvolti non solo alla società calcistica, ma per l'intera economia della città, anche per la socialità, benessere fisico, salute mentale dei cittadini e coesione sociale. Un investimento sulle infrastrutture non si limita allo stadio, ma è un attivatore - come lei diceva giustamente - di altri investimenti su opere pubbliche che mettono in relazione l'impianto con tutta la comunità. Servono stadi più efficienti: lo diciamo da sempre, ma adesso - come lei giustamente ha sottolineato - si sta passando ai fatti. Questi stadi devono essere efficienti anche da un punto vista energetico, quindi coperti e utilizzabili senza limitazioni di tempo per tutto l'anno. È importante quindi, come lei sottolineava, dare unitarietà all'azione in tal senso, proprio in relazione alle attività con le amministrazioni locali e al lavoro che lei sta svolgendo con i club, proprio perché ci sono le condizioni per produrre i fatti, che portino a infrastrutture sportive e arricchiscano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

La seduta è tolta